come lei avrà potuto leggere sulle agenzie e anche sui giornali di oggi, il mio partito oggi pomeriggio si riunirà alle ore 18 per

io credo che debba essere rispettato il travaglio del partito rappresentato dalla senatrice Bianconi.

anzi il dovere di concludere i lavori giovedì con le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, con una intelligente organizzazione dei lavori sarà possibile accogliere la richiesta avanzata dalla senatrice Bianconi.

del quale anche questo provvedimento ha evidente bisogno.

di mantenere l'impegno che l'Assemblea ha assunto - ed è quindi anche responsabilità del Gruppo della senatrice Bianconi accettare che le dinamiche siano queste - da parte nostra non vi è opposizione. Diamo la disponibilità, come abbiamo sempre fatto, ad

Signor Presidente, per un'armonizzazione dei tempi, si potrebbe prevedere la fine dei lavori domani a mezzanotte anziché alle ore 22, e spostare le dichiarazioni di voto dalle ore 11 alle ore 12... Signor Presidente, Senatore Quagliariello, abbiamo già stabilito che alle ore 11 di giovedì inizieranno le dichiarazioni di voto.

La Presidenza purtroppo non può legare o blindare i senatori in Aula. Se dovesse venir meno il numero legale, lei sa che questo non consentirebbe di lavorare negli orari da lei proposti.

Conformemente a quanto già stabilito nel corso dell'esame in Commissione, gli emendamenti da 01.40 a 01.153, a pagina 115 del Tomo I, sono improponibili in quanto volti ad introdurre nell'articolato temi che non formano oggetto del disegno di legge quali il divieto di eutanasia o l'istigazione al suicidio e il riconoscimento e la tutela del diritto alla terapia del dolore, qualificata come finalità esclusiva del disegno di legge. La Presidenza, conformemente a quanto già stabilito nel corso dell'esame in Commissione, dichiara altresì improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti riportati negli elenchi in distribuzione, in quanto estranei al contenuto del disegno di legge in esame, che reca norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Dichiara altresì inammissibili gli emendamenti parimenti riportati negli elenchi in distribuzione in quanto recanti un contenuto manifestamente *ioci causa* o privi di reale portata modificativa.

**Il Senato non approva.**

Presidente, l'emendamento 1.818 propone di aggiungere tra i princìpi costituzionali ai quali il provvedimento che ci accingiamo a votare deve sottostare anche quello di uguaglianza formale e sostanziale: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Ciò, a nostro avviso, deve essere a maggior ragione vero e rispettato quando ci si appresta a intervenire su temi delicati quali la malattia e la vita. Pensiamo, ad esempio, a quanto condizioni di fragilità, marginalità sociale, mancanza di sostegno economico possano influire nelle decisioni sul fine vita. Richiamare il principio di uguaglianza

debba imporre trattamenti non proporzionati o inadeguati o, a quel punto, sostanzialmente inutili. L'emendamento serve a scandire la contrarietà, anche di chi è contrario a questa legge, come si sta facendo, al cosiddetto accanimento terapeutico. Stiamo procedendo in maniera abbastanza rapida in questo avvio d'esame, a dimostrazione che non c'è un intento ostruzionistico. Tuttavia, credo che sarà necessario, man mano che discuteremo, entrare sui punti che stanno a cuore a coloro che hanno svolto un'attività emendativa. Il mio Gruppo, peraltro, ha discusso al proprio interno, nel rispetto di tutte le posizioni, ed è prevalsa un'opinione contraria per una serie di valutazioni di merito e tecniche. Questo è uno dei punti che vogliamo ribadire perché è proprio di chi è contrario a questo tipo di attività legislativa e privilegia la cosiddetta alleanza terapeutica tra medico e paziente nella fase in cui la vita si esaurisce e arriva la morte, quando, quindi, i familiari e i medici sono chiamati

è contrario a questo provvedimento immagina che si debba andare oltre i limiti ragionevoli. Il problema è proprio questo: mettere al bando le pratiche eventuali di accanimento terapeutico non deve portare all'eccesso opposto. Di questo si occupano altri emendamenti circa il ruolo del medico e la sua funzione di tutela della vita, finché di vita si tratta.

non siamo d'accordo, probabilmente e mi riferisco al fatto che negare idratazione e alimentazione possa portare di fatto a un'eutanasia e quindi che l'idratazione e l'alimentazione siano dei medicinali invece che una forma di

estremi da evitare, ad avviso mio e di molti colleghi. Il primo estremo da evitare è pensare che la medicina e la scienza debbano andare oltre qualsiasi limite. Questo non è possibile, benché oggi le cose siano molto cambiate e laddove la terapia, le medicine e i farmaci consentono Grazie avrebbero portato inevitabilmente alla morte del paziente, oggi vengono affrontate e risolte nel giro di ventiquattro ore. Non sono medico e quindi non voglio scendere nel tecnicismo; nell'Assemblea ci sono medici che meglio di me possono illustrare i portenti - almeno, io che non sono medico così li giudico - della scienza medica nel campo

non c'è dubbio che entriamo nell'accanimento terapeutico o addirittura, Dio non voglia, in forme di sperimentazione. Questo emendamento dice di non ricorrere mai all'accanimento, l'uomo non ne ha il diritto. Qui non è un problema di credenti o non credenti: io e credo anche altri colleghi non abbiamo affrontato questo dibattito con un approccio religioso o teologico. Le fedi religiose sono fuori dall'attività legislativa laica di un Parlamento. Il tema del fine vita e di questo confine labile deve essere affrontato in termini legislativi e l'emendamento 1.855 serve a dire che chi è contro questa legge invoca l'alleanza terapeutica e dice che ci vorrebbe un registro. Anche i proponenti di questa legge si sono accorti che è sbagliata, tant'è che vogliono mettere il registro delle DAT

Stefani).* Gli studenti sono andati via, ma ne verranno altri e glielo ridiremo: si sta facendo una modifica alla legge di bilancio che ancora non c'è attraverso la legge di bilancio che ancora non c'è. Questo si sta facendo. È una tecnica legislativa corretta?

una forma di accanimento legislativo, per cui mi accorgo dell'errore ma non lo cambio perché siamo a fine legislatura (non a fine vita), lo metto nella legge di bilancio, mi rimbalza qui la legge e non si capisce più niente. Non è che un registro sia una cosa banale,

credo si possa ritenere che gli emendamenti 1.858 e 1.859 contengano il cuore delle ragioni divisive che si sono sin qui manifestate. Infatti, tali emendamenti vorrebbero sopprimere il concetto di autodeterminazione, riferito, oltre tutto, ad una situazione futura e, quindi, non un'autodeterminazione che si esprime in una condizione attuale e concreta.

Grazie Questo è il tema che più oppone i due schieramenti che si sono confrontati con riferimento al provvedimento Sarebbe invece utile un ascolto reciproco e la ricerca di un punto di compromesso a questo proposito. Voglio soprattutto segnalare che l'affermazione dell'autodeterminazione assoluta del paziente combinata oltretutto con un registro fragile, come quello cui poco fa ha fatto riferimento il collega Gasparri, determinerà ragionevolmente l'inibizione di molti medici, chiamati a rianimare un paziente, ad attendere non solo la ricerca di eventuali dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, ma in ogni caso anche a temere un'attività rianimatoria dalla quale potrebbe derivare, malauguratamente, l'esito di una

del Servizio sanitario e, in generale, l'orientamento alla vita della professione medica, già sottoposta a frequenti azioni di responsabilità civile. Qui come altrove, insomma, rivolgiamo davvero un appello alla ricerca di una sintesi. Mi rendo conto che, probabilmente, non ve ne sono qui le condizioni, data l'assoluta determinazione con cui si vuole approvare questo provvedimento, anche in assenza di soluzioni all'evidente carenza di pubblicità e di certezza della dichiarazione anticipata di trattamento, anche in presenza, cioè, di un vuoto normativo che si vuole colmare confusamente, nei termini ricordati da Gasparri poco fa, attraverso la legge di bilancio.

lasciano dietro di sé effetti devastanti. Credo nella società e nelle stesse funzioni pubbliche dedicate alla salute. Mi auguro solo che un Parlamento diverso possa avere la saggezza che questo Parlamento sembra non avere, nemmeno a questo proposito.

il trattamento da utilizzare con i minori, nel caso, per esempio, di contrasto tra i medici curanti e gli affidatari. Ricordo il precedente giurisprudenziale di Luana Englaro.

tuttavia una vita affidata alle cure amorose delle suore: la alzavano, la vestivano, la portavano fuori, le facevano prendere il sole. Quindi, era all'interno di una specie di placenta dove viveva una sua vita protetta. Bene, anzi male: da questa sua vita protetta è stata scaraventata su un'ambulanza che l'ha portata a centinaia di chilometri lontano: l'hanno messa in una stanza dove, non dandole più alimentazione, in qualche giorno è morta nella maniera Grazie Come ho detto in discussione generale, non credo sia stato un gran progresso per Luana lasciare la sua vita, ripeto, anche se vegetale: anche una pianta non la si fa morire non dandole da bere e facendola seccare. Sarebbe contro la coscienza comune arrivare a soluzioni così crudeli.

ci sono personale specializzato e volontari che seguono bambini che non hanno alcuna possibilità di guarigione,

volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia. I bambini sono incapaci d'intendere e volere. Quindi, con questo emendamento si dice che questi bambini hanno diritto di avere un sostegno.

deve smettere di essere alimentato e deve morire? Che cosa succede? L'articolo 4 una risposta la dà: è il magistrato che decide. È esattamente il caso di Charlie Gard, che ha commosso e indignato tutto il mondo, perché in quel caso erano i genitori a dire: vogliamo continuare le cure per nostro figlio, perché finché c'è vita c'è speranza, perché esistono terapie innovative, ma il magistrato lo ha condannato a morire. a morire. Vorrei che qualcuno dei colleghi della maggioranza mi spiegasse se ciò che ho detto non corrisponde a verità storicamente, con il caso di Eluana, e se, in prospettiva, le norme che andiamo ad approvare non si debbano applicare invece a centinaia di casi. Non stiamo parlando di persone che, essendo coscienti e maggiorenni, decidono di non avvalersi delle cure, come già in Italia avviene. Non parliamo di persone, maggiorenni,

di persone alle quali si applicano queste regole e queste leggi senza che loro siano mai state in grado di esprimere la loro volontà. Faremo un salto di civiltà nel senso che a questi bambini verrà negata la possibilità di vivere la loro vita? Ci sarà qualcuno che stabilirà quando la vita sarà degna o no di essere vissuta? Ci sarà qualche tribunale che stabilirà che quei bambini devono morire sotto forma di interruzione dell'alimentazione e del sostegno vitale? Io voglio delle risposte a queste domande perché, come ha detto prima il collega Sacconi, per i bambini c'è questo problema, ma per gli adulti non c'è un problema minore.

sulla base di quello che c'è scritto e c'è scritto esattamente questo, e non altro. Questo prevede il provvedimento. Lo prevede per i minori e poi lo richiama nel confronto che c'è fra l'affidatario e il medico quando discutono per le DAT.

prima di intervenire. Certo, dovrà andare a scartabellare in tutte le Regioni d'Italia perché, non essendovi un registro nazionale, nessuno è in grado di sapere in tempo reale la volontà di colui che viene ricoverato.

e «garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere», cioè dei minori, questa è una scelta di civiltà, non quella di abbandonarli. Quindi, io voterò decisamente a favore di questo emendamento. Presidente, intervengo per supportare l'emendamento 1.858 e per confermare quanto diciamo da tempo e che abbiamo detto anche durante la discussione generale. Noi chiediamo la soppressione della parola autodeterminazione per il semplice motivo che sappiamo benissimo che nella filosofia sottesa a questo argomento ci sono due modi di pensare, come abbiamo detto anche in discussione generale: un modo di pensare che parla della autodeterminazione della propria vita, quello che state portando avanti voi, e un altro modo di pensare, che è il nostro, che è quello della inviolabilità della vita. Il problema, colleghi, è che tutti sanno che quando si parla di autodeterminazione della propria vita, la direzione, la conseguenza, il punto di arrivo è il suicidio assistito e l'eutanasia ed è per questo motivo che avete dichiarato inammissibili tutti i nostri emendamenti quando si parlava di eutanasia. Questa è una legge che porta all'eutanasia, lo abbiamo detto in tutte le lingue e andremo avanti a dirlo in tutte le lingue, e la parola autodeterminazione è la conferma di quello che stiamo dicendo. Presidente, chiedo scusa a tutti coloro i quali non la pensano come me, però dagli interventi che abbiamo sentito si capisce perfettamente che la costrizione a sospendere l'idratazione e l'alimentazione, se assistite, accompagnata da un trattamento di sedazione profonda, significa eutanasia.

appartenenza. Faccio questa riflessione perché mi sento in grande difficoltà e non so se effettivamente, in questo momento, sto assumendo

del vice presidente Gasparri, ma per avere un aiuto a comprendere): la libertà di coscienza all'interno di quest'Aula, che significa? Io che appartengo ad una cultura, posso rinnegare questa mia cultura, posso rinnegare il mio Dio in un momento difficile cui devo dare anche conto alla mia coscienza? Posso dire, in questo preciso istante, che la mia libertà di coscienza mi libera dal dover votare contro un mio credo? Posso votare l'eutanasia nascosta attraverso Signor Presidente, chiedo scusa a tutti coloro i quali non la pensano come me, ma questo è un argomento delicato e io ho necessità di interrogarmi, alla presenza non di coloro i quali non credono e sono atei, ma alla presenza di coloro i quali credono e sono di coloro i quali credono e sono credenti all'interno di quest'Aula e mi devono spiegare che cosa significa libertà di coscienza: significa votare senza alcun riferimento al proprio credo, alla propria dottrina ed alla propria cultura, oppure significa votare in votare in rapporto al proprio credo e alle proprie radici di appartenenza? Quando allora oggi si propone non con chiarezza, signor Presidente, di votare una di votare una legge che porta alla legittimazione dell'eutanasia, possiamo noi fare finta di non vedere, di non capire e votarla? No, non possiamo farlo, perché una cosa è parlare di quello che abbiamo messo all'ordine del giorno, un'altra cosa è parlare senza distinguere verità e falsità. La falsità non ci appartiene per cultura: a noi appartiene la verità. Su questo argomento c'è un problema delicatissimo, che non investe solo ed esclusivamente ciò che noi delibereremo oggi, ma ciò che sarà il futuro per noi, per i nostri figli e per i nostri nipoti.

di essere cattolici, ortodossi, evangelisti, perfettamente convinti e credenti. PRESIDENTE.

come mai la maggioranza del Senato vota contro princìpi costituzionali e lo stesso Governo si rimette all'Assemblea? Anche noi votiamo alcune cose sbagliate. In questo emendamento c'è un principio sacrosanto che legittima la spiegazione dei princìpi già affermati nel disegno di legge. Ma qui era necessario un intervento del Governo. Non bisogna togliere la togliere la parola «autodeterminazione», che rientra nei princìpi costituzionali; bisogna scrivere garantendo politiche sociali ed economiche agli handicappati e agli incapaci:

istituzionale e chiarendo il senso delle parole. L'autodeterminazione non significa nulla se poi non è garantita a chi non ha autodeterminazione perché

Da una parte si vota contro, dall'altra si vota a favore, ma senza un minimo di dibattito, di dialogo e di spiegazione delle ragioni per cui si vota contro.

Signor Presidente, a differenza di altri colleghi io non credo che il problema in quest'Assemblea sia la divisione tra chi crede e chi non crede. A dimostrazione di ciò vi sono stati tanti colleghi che, a sostegno del disegno di legge in esame, hanno detto che non ha nulla a che vedere con il diritto all'eutanasia.

di questo provvedimento, hanno affermato che esso non reca il diritto all'eutanasia ma la via italiana all'eutanasia, cioè apre degli spiragli all'interno dei quali

la distinzione e consentire a quanti ritengono che una legge sulle DAT sia assolutamente legittima, in quanto

un principio chiaro per cui non vi può essere alcun diritto di autodeterminazione della persona che si spinga fino a violare il principio di inviolabilità e indisponibilità Per questo si propone di richiamare apertamente gli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e di esplicitare il divieto a qualsiasi forma di eutanasia e di assistenza al suicidio. Si afferma inoltre che l'attività medica non può essere che esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della

a questa normativa e fissiamo anche il fatto che il medico debba astenersi da trattamenti straordinari e non proporzionati, ovvero da qualsiasi forma di accanimento terapeutico. Se lo scopo è rafforzare il divieto all'accanimento terapeutico e tener conto della sofferenza,

prendere veramente in carico i pazienti. Un compito della società civile è tutelare la vita dei cittadini, assicurando loro tutti i mezzi a disposizione per le terapie curative o palliative migliori, e garantire un'esistenza dignitosa fino alla morte. Attualmente lo Stato non lo fa. Abbiamo visto cos'è stato dato per il *caregiver* familiare: praticamente alle famiglie dei disabili arrivano circa 7 euro l'anno. È veramente vergognoso, una presa in giro. Lo scopo di questo emendamento è evitare casi strazianti come quello del disabile che è dovuto andare in Svizzera a chiedere l'eutanasia perché lo Stato non lo prendeva in carico secondo i suoi diritti umani e costituzionali.

Il Parlamento sembra accingersi ad approvare questa soluzione nel segno dello scarto Grazie Grazie e di un decreto ministeriale del 2015 sui parametri minimi di efficienza delle strutture sanitarie. Avremmo il dovere di chiudere territori ospedali marginali - sono circa 200 - che costituiscono un'immanente pericolo per le persone che, in uno stato di bisogno acuto, vi vengono ricoverate. La loro chiusura non determinerebbe solo economie riferite ai costi fissi, ma soprattutto determinerebbe un minore ricorso a ricoveri inappropriati, perché l'eccesso di offerta, soprattutto di offerta di offerta marginale, tende ad attrarre e accrescere la domanda. Queste risorse si rivolgerebbero invece ai servizi territoriali, a sostegno delle cure domiciliari in modo particolare, o in ogni caso a sostegno della domanda delle persone che si trovano in condizione di bisogno cronico. Dovremmo quindi realizzare quelle proporzioni tra i macrolivelli di assistenza, che definimmo costi *standard* in occasione della legge sul federalismo fiscale, che lei Presidente ricorda bene e che prevedevano la spesa per spedalità al 44 per cento, la spesa per prevenzione al 5 e una spesa maggioritaria in ciascun ambito territoriale proprio per quei servizi che sono rivolti a trattare appropriatamente in particolare le persone in condizioni di disabilità, soprattutto laddove la famiglia voglia

essere salvata attraverso il ruolo responsabile, in scienza e coscienza, del medico, tramite quel parametro che, con una parola, potremmo chiamare appropriatezza, che invece qui verrà meno, irrigidendo tutti i comportamenti della professione medica e sovvertendo tutto l'impianto del servizio sanitario nazionale, sin qui orientato alla vita. non mi sembra che l'emendamento della senatrice Rizzotti sia irrilevante. esso rientra nella tipologia di quegli emendamenti che vorrebbero espellere dal testo il principio di autodeterminazione. Nello stesso tempo, però, è un emendamento che ci dimostra quanto abusivamente la categoria dell'autodeterminazione sia diventata di una latitudine sterminata nel Qualche minuto fa il senatore Caliendo ha richiamato, ai fini di un corretto lavoro legislativo,

che se prevalesse, ma nella latitudine dell'autodeterminazione, la categoria dello scarto, allora, in termini di politica sociale,

il Governo, per coprire un legislatore amico che ha preso la categoria dell'autodeterminazione e l'ha dilatata al massimo dei massimi, essere insensibile al proprio diritto-dovere di chiarire gli aspetti sociali di questa scelta. Del resto, signor Presidente, su che cosa si era

il ruolo del medico, che qui è furbescamente incardinato nella libertà di autodeterminazione.

allora è soltanto cinismo invocare questa larghezza di autodeterminazione. L'autodeterminazione

chi è che decide? Da lui viene rivendicato il massimo dei sovranismi, nel senso della libertà individuale (non siamo sul terreno del diritto costituzionale). Francamente io non l'ho mai pensata come lui, anche quando ero nella condizione di paziente, infartuato, non so se consapevole o quanto inconsapevole; non ho mai preteso di decidere io: decidessero mia moglie, i miei figli, il medico. Questa è l'alleanza terapeutica. Questa volgare dilatazione dell'autodeterminazione ci porta all'assurdo. L'avete negato negli emendamenti precedenti, ma una sinistra che ha una cultura dello Stato sociale come fa a non aver niente da dire sulle implicazioni dell'emendamento della collega Rizzotti?

introduce una precisazione importante, altrimenti il testo che abbiamo di fronte direbbe che la presente legge «stabilisce che

che, per suoi motivi di forte convincimento, vuole effettivamente darsi la morte o lasciarsi morire in quella certa situazione. Chiunque, spinto sia da un obbligo, innanzitutto, credo, morale, sia dagli obblighi di legge (perché ricordo che l'omissione di soccorso è reato),

L'urgenza è tutt'altro che un caso strano in medicina: i reparti di pronto soccorso a cosa servono? Pertanto mi sembra doverosa l'approvazione di questo emendamento. finestra"). Comunico che è pervenuta una richiesta di votazione con scrutinio segreto. riterrà accoglibile tale richiesta rispetto a emendamenti che verranno votati nella seduta successiva a quella odierna, non avendo il tempo materiale per poter valutare l'accoglibilità

Grazie

Grazie tutti gli emendamenti o quelle parti di essi che vietano il ricorso a pratiche eutanasiche. Poiché per molti di noi in questa Aula valgono i due paletti del rifiuto dell'accanimento terapeutico, da un lato, e il rifiuto delle pratiche eutanasiche, dall'altro, vorrei comprendere vorrei comprendere - ma penso d'interpretare l'opinione di altri colleghi - la ragione per cui la Presidenza ritiene non votabili tutti i contenuti che esplicitamente proibiscono le pratiche riconducentisi al termine di eutanasia. Senatore Sacconi, la stessa eccezione è stata sollevata dal presidente Centinaio e la risposta rimane la medesima. È valso lo stesso criterio della Commissione e, in più, sono stati illustrati, quando ho dichiarato l'inammissibilità, anche le motivazioni che le hanno determinate.

sono dedicati all'alleanza terapeutica, alla coalizione e cooperazione tra paziente, quando cosciente, i suoi familiari e, soprattutto, il medico che in scienza e coscienza valuta l'appropriatezza delle terapie e delle stesse cure della persona. La ragione principale del dissenso che noi esprimiamo Ricordo ancora una volta, e insisterò quanto più possibile su questa discussione, i pericoli che si determineranno anche per coloro che non presenteranno la Dichiarazione anticipata di trattamento. Ogni medico Ogni medico non potrà che fermarsi di fronte alle proprie convinzioni, di fronte anche a ciò che il suo giuramento, la sua scienza e la sua coscienza gli imporrebbero di fare,

anche con tutta la preoccupazione delle possibili conseguenze di un esito negativo dell'attività di rianimazione. È qui messo in discussione un profilo fondamentale di tutto il nostro Servizio sanitario nazionale; dobbiamo essere consapevoli che qui non si dispone soltanto la possibilità per una persona di rinunciare anticipatamente a determinati trattamenti,

nella nostra esperienza, oltre che nelle nostre leggi e negli statuti che regolano le aziende sanitarie o sociosanitarie. Qui si mette in discussione la la funzione del medico e l'orientamento del servizio sanitario alla vita. La preoccupazione che sorge è legittima e riguarda tutti; anche coloro, i molti, moltissimi che non produrranno una dichiarazione anticipata di trattamento. La preoccupazione è però più in generale rivolta ad una società che, nel momento in cui perderà il senso ed il valore della vita, inesorabilmente accelererà il proprio percorso di declino.

porta in sé una serie di problemi che ne certificano l'inadeguatezza. Nel precedente intervento ho sottolineato come gli stessi sostenitori della legge ne riconoscano gli errori e i limiti proponendo il registro sulle Dichiarazioni anticipate

la negazione dell'obiezione di coscienza, quindi si obbliga il medico a comportamenti che potrebbero legittimamente confliggere con la sua coscienza. Ma come? Si fa appello in tutti i campi, giustamente, alla libertà di coscienza, alla libertà che gli stessi parlamentari su materie come queste devono avere, e poi si nega per legge la libertà di coscienza al medico. Già questo è un modo sbagliato e incostituzionale di legiferare, che porterà a contestazioni quando i medici, anche di fronte a una discussione su singoli casi,

la sua attività di medico, che è un'attività non comune visto che da questa dipendono i destini di ciascuno di noi quando ci si affida in qualsiasi fase alle cure, alle terapie e alle mani - in caso di operazioni - di un medico. Con questa proposta, quindi, richiamiamo un fatto fondamentale. che il ruolo del medico venga strattonato da questo disegno di legge lo conferma anche il fatto che all'articolo 1, comma 6, si stabilisce una sorta di esenzione del medico da responsabilità civili e penali.

Una legge esenta un medico che ha la responsabilità delle scelte; di fronte ai casi concreti è la legge a dire che quello è esente da responsabilità. Insomma, entriamo in una sfera veramente complicata, discutibile e opinabile. senatore Scilipoti Isgrò giustamente richiamava anche altri tipi di dimensione della riflessione, ma io non li evoco, senatore Scilipoti Isgrò, per evitare di rafforzare con altre motivazioni queste argomentazioni. Mi attengo a discorsi proprio di natura medica, scientifica, sanitaria e di tutela della vita, che è un tema che non deve essere solo dei credenti ma di tutti. Io sono credente, però ritengo che anche sui temi fondamentali della vita - come nasce e come finisce - e della genitorialità. Ne discutemmo in altre occasioni su altri provvedimenti: come nasce un bambino e qual è la genesi fisica della nascita. nascita. Il diritto naturale si chiama tale perché riprende dalla natura ciò che avviene secondo princìpi naturali; non è certo la legge a decidere come nascono i bambini. Qualcuno pensa che anche questo si debba fare.

Io stesso, che sono contrario a questo provvedimento, tengo conto di motivazioni emerse - anche diverse da quelle che porto avanti io - che con altri colleghi abbiamo registrato essere prevalenti nel nostro Gruppo. Quando prima ho parlato dell'emendamento contro l'accanimento terapeutico, che avete respinto, ho sostenuto un principio che dovrebbero difendere coloro che vogliono questa legge e che quindi dicono che, a un a un certo punto, la vita va via. Anche lì c'è una contraddizione: di fatto non volete che si scandisca un no più preciso all'accanimento terapeutico, che chi è contro questa legge, sotto altri profili, invece, ritiene di mettere al bando. In questi emendamenti, che certamente non approverete, si parla del consenso informato, della relazione di cura, del rapporto tra paziente e medico e anche di una relazione in cui sono coinvolti i familiari e un eventuale fiduciario. Credo che su questi temi ci

il crinale dell'esaurirsi del rapporto tra vita e morte è quello. Prima avete anche respinto un altro emendamento che la senatrice Rizzotti aveva presentato citando Convenzioni internazionali in cui si precisa che l'idratazione e il nutrimento non sono procedure mediche, ma devono essere somministrate fino a quando possono attivare reazioni fisiologiche (è ovvio, poi, che a un certo punto anche quella fase si esaurisce).

alle Convenzioni internazionali e ai deliberati della scienza, gli scientisti per eccellenza dovrebbero, più di noi, uniformarsi ai princìpi della scienza, che sono una dimensione del sapere umano e della decisione umana, non l'unica per tutti, ma certamente sono un aspetto importante. Qui voi state votando anche contro la scienza, contro la scienza medica e contro le deliberazioni delle organizzazioni internazionali. L'oscurantismo, che a volte viene attribuito a chi contrasta questa legge, è proprio di chi, in maniera ideologica, apodittica e pregiudiziale,

saranno medici e operatori della sanità, infatti, a contestare l'incostituzionalità dell'obbligo eutanasico che deriva da queste legge. E nessuna legge, cari colleghi, potrà trasformare in potenziali omicidi dei medici che non volessero aderire a questo principio legislativo: si richiameranno alla Costituzione, ai princìpi fondamentali, e poi

di chi fa osservazioni motivate, non ideologiche, ma sicuramente più scientifiche degli anti-scientisti che bocciano anche le Convenzioni internazionali sull'idratazione e sul nutrimento.

di alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. I nostri emendamenti sono di buon senso: qui non c'è niente di politico, di ostruzionistico, di tecnicamente non condivisibile; sono tutti emendamenti di buon senso. Sono emendamenti che potrebbero essere approvati

in esame con cui si autorizzerà l'eutanasia, si toglie invece anche quella destinazione e quell'*input* che si dà alla professione medica: quella di cercare di salvare la vita. Questo emendamento va in quella direzione. Noi siamo dell'idea di votare a favore,

Signor Presidente, intervengo anche sull'emendamento 1.973. Questi emendamenti mirano a reinquadrare correttamente il tema del consenso informato

l'atto fondante dell'alleanza terapeutica è stato spesso ridotto a mero atto burocratico funzionale, più che altro serve ad offrire una tutela al medico rispetto a eventuali e futuri contenziosi. Questa lettura del consenso informato è riduttiva e fuorviante, perché il consenso informato deve essere a monte della relazione tra medico e paziente, che deve invece divenire una vera e propria alleanza terapeutica e non, come questa legge vorrebbe, un mero atto legale e burocratico fatto solo di moduli da leggere e da compilare. Signor Presidente, questi due emendamenti provano a reinquadrare questo punto fondamentale e a farne un atto vero e vivo, sottraendolo alla burocrazia.

Signor Presidente, intervengo anche sul successivo emendamento 1.5005, perché questi due emendamenti fondano la propria ragion d'essere su una corretta definizione del rapporto tra medico e paziente, la cosiddetta alleanza terapeutica, che deve determinarsi nel processo di redazione delle DAT. In particolare, ciò è motivato dal fatto che anche in una situazione estrema in cui il soggetto, cioè il paziente, non è più in grado di esprimersi, il rapporto di fiducia che lo lega al suo medico - a volte sin dalla si concretizza nel dovere del medico di prestare tutte le cure di fine vita, agendo sempre nell'interesse esclusivo del bene del paziente. Non si può non tenere in debita considerazione che le dichiarazioni anticipate di trattamento sono sicuramente espressione della libertà del soggetto di esprimere i propri orientamenti circa i trattamenti sanitari cui deve essere sottoposto nell'eventualità di trovarsi in condizioni di incapacità di intendere e di volere ma, allo stesso tempo, lo privano della possibilità di contestualizzare e di attualizzare la sua scelta. Il diritto di autodeterminazione, per non divenire costrizione tirannica su se stesso, deve sempre lasciare uno spiraglio alla revisione e persino alla contraddizione. Questo è vero soprattutto quando la persona si riferisce ad uno stato che non conosce, di cui non ha avuto esperienza. Noi sappiamo che la libertà deriva anche da un dato di esperienza effettivo. In caso contrario, se di questo dato di esperienza non si tiene conto, la libertà si trasforma in quella che è stata opportunamente definita da alcuni filosofi «presunzione fatale»; presunzione fatale di poter determinare il proprio destino una volta per tutte, senza tenere conto dei mutamenti, delle trasformazioni, delle sorprese, della meraviglia che la vita sa riservare ogni giorno. Questa concezione di libertà aperta all'empiria e alla relazione, e per questo mai assoluta, interpreta, signor Presidente, un'idea di laicità comune a credenti e non credenti. Se è vero che per un credente la vita è aperta a qualsiasi determinazione fino in fondo, è altrettanto vero che per un laico liberale il futuro è aperto per definizione; se lo si chiude, se lo si lega a una dichiarazione anticipata, magari anche di molti anni, in realtà si finisce per contraddire l'idea stessa di libertà. Con questi due emendamenti Con questi due emendamenti abbiamo inteso che il concetto di alleanza terapeutica rappresenti la possibile traduzione di questa concezione della libertà, conferendo al paziente l'autonomia di orientare le sue scelte terapeutiche in un contesto per lui ignoto, e al medico la responsabilità, nella situazione data, di attualizzarne le indicazioni. In questo contesto, il medico può assumere in maniera corretta le decisioni più opportune per il paziente, tenendo conto attentamente attentamente della sua volontà alla luce di nuove circostanze che si sono eventualmente venute a creare e sempre in applicazione del principio della tutela della salute e della vita umana, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità Signor Presidente, visto che gli emendamenti - diciamo così - sul divieto di eutanasia sono caduti, questa concezione della libertà del paziente e della responsabilità del medico traducono, a nostro avviso, l'esatto confine che passa tra l'esplicazione di dichiarazioni anticipate di volontà e invece una concezione più rigida che, per forza di cose,

quando ci saranno emendamenti nell'ambito dei quali vorrei intervenire. Grazie ancora. intervengo a proposito di questi emendamenti e di quelli successivi, tra i quali uno a mia prima firma, l'emendamento 1.982, sempre con riferimento al rapporto tra medico e paziente; rapporto che, pur dovendo necessariamente basarsi sulla fiducia e sul rispetto reciproci, non potrà mai essere simmetrico. È infatti il paziente che si affida al medico e non viceversa, mentre è il medico che ha una precisa responsabilità nei confronti del paziente, conformemente al codice deontologico. caso invece si determina addirittura una asimmetria rovesciata: è il paziente che esprime anticipatamente un ordine vincolante ed il medico è chiamato ad eseguirlo ed è proprio su questo punto, come ha detto poco fa il collega Quagliariello, che si consuma il confine che ci conduce all'eutanasia.

ravvisano significativi elementi che conducono a pratiche eutanasiche; non ci è però consentito di esprimere un voto esplicitamente contrario ad esse, in modo da definire un paletto non superabile, quello proprio dell'eutanasia. Si è detto molto fuori di queste Aule, anche autorevolmente, che occorre evitare tanto l'accanimento terapeutico quanto l'eutanasia, ma qui dentro non ci è consentito esprimere un voto Grazie Quando il medico si riduce a mero esecutore, quando nella sua attività lo si priva di ogni riferimento a codici deontologici,

Presidente, siamo su uno dei punti fondamentali del dibattito che noi vogliamo richiamare e sottolineare. Abbiamo già parlato di tutto ciò che avviene nel campo della professione medica.

In questo caso riteniamo che il concetto dell'alleanza terapeutica - lo vogliamo ribadire - sia il fondamento vero delle decisioni da assumere. prima, ognuno di noi nella vita ha avuto un'esperienza in cui si esaurisce la vita di un congiunto o di un parente e in cui il medico a un certo punto ci ha messo di fronte all'amara realtà, dopo le cure e dopo tutto quello che viene fatto.

possono fare delle valutazioni sotto il profilo medico, sanitario, della qualità di vita, dell'efficacia o meno dell'idratazione e del nutrimento, che quando non sono più in grado di attivare processi fisiologici non hanno più senso neanche loro. quindi un furore ideologico che nasconde una volontà - poi quando lo diciamo qualcuno si arrabbia - di introdurre un principio di eutanasia. Tanto è vero che poi al medico si dice che non sarà responsabile penalmente e civilmente. Chi l'ha detto? E dove si decide? Poi ci sarà una legge che verrà superata da un'altra legge; ci sarà un principio costituzionale che sarà invocato dalla coscienza del medico. Stiamo quindi facendo una legge che entra in sfere molto delicate e complesse e che apre un contenzioso, perché non c'è solo il contenzioso che qualcuno ha aperto in passato, ottenendo pronunciamenti della Cassazione che sono stati arbitrariamente interpretati, visto che anche su casi eclatanti che nel passato hanno scandito la vita italiana e anche la vita di questa Assemblea del Senato ci sarebbe molto da dire: sentenze che non erano sentenze e pronunciamenti che non erano pronunciamenti. Leggi fatte male aprono la strada a sentenze fatte peggio e a incertezze ancora maggiori. Solo che stiamo parlando della vita e della morte delle persone. È allora molto meglio richiamarsi all'alleanza terapeutica tra chi ha la competenza - nel caso del medico - e i familiari e le altre persone che possono assumere decisioni curative che non questa normativa che aprirà la strada all'eutanasia; poi arriverà qualche sentenza, poi qualche contestazione e poi, com'è successo per altre materie altrettanto rilevanti e delicate, andrà tutto davanti alla Corte costituzionale che forse "praticherà l'eutanasia" su una legge sbagliata, in quel caso agendo legittimamente. Quindi vi invitiamo a votare a favore del principio dell'alleanza terapeutica per affidare al buon senso, alla competenza, alla scienza e alla coscienza di medici e familiari le decisioni che vanno prese, invece che imporre con una legge delle norme che vanno contro il codice penale, tant'è che si dice: chi lo farà, non è colpevole. Si sa già, evidentemente, che non tutto quadra. Legiferare così così è molto sbagliato, cari studenti. So che non bisogna rivolgersi agli studenti, ma alla Presidenza, ma oltre a fare la visita, in questo modo approfondiscono anche le modalità con cui si fanno le leggi e queste sono molto discutibili e sbagliate, come metodo prima ancora che nel merito, caro Presidente.

si è guastato. Questo è un messaggio subliminale del sistema di votazione elettorale per indurci a più miti consigli.

Avverto che, conformemente alle determinazioni adottate dalla Conferenza dei Capigruppo di martedì 5 dicembre 2017, dopo le comunicazioni si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulle proposte di risoluzione presentate.

degli anni, le comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo

binario tra temi particolari, sui quali il Consiglio europeo deciderà, e temi molto generali, sui quali proseguirà o avvierà il confronto.

ci sono stati il risultato del *referendum* britannico e, per certi versi, anche il risultato delle elezioni americane, che hanno configurato in un modo diverso i rapporti tra l'Europa e il suo storico e attuale principale alleato. Si potrebbe poi dire che il 2017 è stato l'anno della risposta a questo doppio *shock*, di una ripresa di speranza e di impegno dal punto di vista dello slancio europeista, con alcune decisioni, incontri e con alcuni risultati elettorali. Adesso siamo alla vigilia del 2018: un anno che può rivelarsi decisivo perché alla fine si vedrà se, dal risveglio europeista di cui siamo stati testimoni nelle forme più diverse nel corso dell'anno che sta terminando, si passerà a una fase di passi concreti in direzione dell'attuazione di alcune delle dichiarazioni, delle ispirazioni e dei progetti che si sono sentiti in questi mesi; oppure se saremo condannati un po' a un anno di *surplus*, a causa della durata, più lunga del previsto, del negoziato per la formazione del nuovo Governo tedesco, nonché a causa dell'attesa per le elezioni nel nostro Paese Paese o, in generale, per mancanza di determinazione, di coraggio e di unità da parte dei Governi europei. Credo che l'Italia abbia tutto l'interesse a evitare questo rischio, a evitare cioè il rischio di un 2018 in cui le prospettive, gli orizzonti e le ambizioni che si sono manifestati negli ultimi mesi finiscano per essere delusi. E, quindi, è importante che si vada a queste discussioni con propositi e idee piuttosto chiari, risoluti e definiti. Faccio un passo indietro semplicemente per informare il Senato dei temi, per quanto circoscritti, sui quali si prenderanno delle decisioni, prima di passare a quelli più strategici ai quali l'Italia porterà le posizioni del nostro Paese. La decisione principale riguarderà, nella giornata di venerdì, la presa d'atto dei risultati che consideriamo positivi della prima fase del negoziato con il Governo britannico. Un anno dopo la scelta del *referendum,* la decisione a maggioranza, che ovviamente abbiamo sempre considerato con rispetto, dell'elettorato del Regno Unito di uscire dall'Unione europea è stata certamente uno *shock* per noi, ma ha creato problemi molto rilevanti da ogni punto di vista, politico ed economico - certamente noi non abbiamo alcun compiacimento nel registrarli - allo stesso Regno Unito. Era l'apice di una fase di crisi. È stata in fondo una sveglia per l'Unione europea

dall'esito del *referendum* britannico e da ciò che è capitato al Regno Unito dopo il *referendum* ci sia stata una grande disseminazione di posizioni antieuropee e vogliose di imitare quella soluzione e quel risultato. Al contrario, oggi ci sono difficoltà evidenti nel Regno Unito, alle quali dobbiamo guardare con il rispetto che si deve a un Paese amico e alleato dell'Italia in tantissime occasioni della storia recente e, tuttavia, constatando che la scelta di uscire è stata veramente difficile. I negoziati hanno raggiunto progressi sufficienti. E ciò verrà sancito dal Consiglio europeo nella giornata di venerdì nei tre *dossier* che erano all'ordine del giorno di questa prima fase, come già sapete. i rapporti con la questione irlandese. Sarebbe stato molto pericoloso che l'uscita dall'Unione europea riaccendesse la questione irlandese. a una definizione per la quale non ci saranno controlli di confine né tra Belfast e Dublino, né tra Belfast e Londra. Non sarà facile tradurre questa scelta in pratiche concrete, ma credo sia un risultato importante. In secondo luogo, si è risolta la discussione forse più difficile per l'opinione pubblica britannica sull'ammontare delle somme dovute dal Regno Unito al bilancio europeo. E si è risolta con piena soddisfazione dei negoziatori dell'Unione europea perché - senza entrare nel dettaglio delle cifre - si è riconosciuto l'impegno da parte britannica di corrispondere tutto ciò che è dovuto al bilancio europeo, inclusi la Banca europea degli investimenti e altre agenzie con alcune limitatissime eccezioni, sulle quali la discussione continua. In terzo luogo - è la cosa che forse interessa di più una parte dei nostri connazionali, alcune centinaia di migliaia di italiani che vivono nel Regno Unito - si è risolta la questione dello *status* dei cittadini comunitari che risiedono nel Regno Unito, riconoscendone i diritti acquisiti e anche dichiarando una volontà da parte del Governo di Londra di rendere il più facile possibile la transizione da uno*status* all'altro. Ci sarà, quindi, la conversione automatica degli attuali documenti di residenza nei nuovi certificati; uno dei punti apparentemente marginali, ma più rilevanti della discussione. Anche a tal riguardo ci sono alcuni aspetti secondari ancora in discussione, ma credo verranno risolti. Dobbiamo tuttavia essere consapevoli che la seconda fase del negoziato con Londra non sarà più semplice, ma più complicata della prima fase. della prima fase. Come sempre, i divorzi sono più difficili dei matrimoni e, in questo caso, è evidente che definire le relazioni tra l'Unione e il Regno Unito diventato Paese terzo sarà un'operazione molto complessa dal punto di vista giuridico, tecnico, economico e amministrativo. Credo che noi italiani dobbiamo predisporci a questo esercizio con l'atteggiamento di amicizia che abbiamo sempre avuto, difendendo i nostri interessi nazionali, ma sapendo che la strada del *no deal*, di non trovare un accordo e lasciare tutto alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio, sarebbe un ripiego negativo e pericoloso. È quindi nell'interesse dell'Europa e del nostro Paese arrivare a un'intesa. di un'intesa che molto probabilmente avrà due fasi distinte: una fase di transizione, di un paio di anni, dalla data fatidica del 29 marzo 2019, in cui avverrà la separazione del Regno Unito dall'Unione europea e, poi, vi sarà un nuovo regime di rapporti tra l'Unione e il Regno Unito. bene comunque che la prima fase si sia conclusa con soddisfazione da parte dei negoziatori europei e con un grado di unità dei 27 Paesi dell'Unione assolutamente rimarchevole. Se qualcuno quindi pensava di poter gestire questo negoziato facendo leva su divisioni tra i Paesi dell'Unione europea, ha sbagliato i propri conti e, da questo punto di vista, l'atteggiamento è molto positivo. le altre due decisioni che verranno prese nel Consiglio europeo, la prima concerne il settore della difesa, la cooperazione rafforzata nel campo della difesa e il varo di alcuni progetti industriali di difesa comune. Sarà una decisione in qualche modo solennizzata dal Consiglio europeo. Se dicessi che è una decisione di per sé all'altezza della domanda geopolitica di Europa che c'è in questo momento nel mondo, obiettivamente andrei un po' al di là della realtà di queste decisioni. Stiamo sempre parlando di primi passi, sia pur positivi e incoraggianti; incoraggianti soprattutto da due punti di vista. In primo luogo si parla di progetti industriali comuni. comuni. Noi ci stiamo portando avanti su alcune materie, e penso - ad esempio - alla cantieristica e all'accordo che abbiamo fatto alcuni mesi fa.

non tutti i 27 o 28 dell'Unione europea. È una prima e significativa traduzione in pratica di un principio che abbiamo affermato nella dichiarazione di Roma del marzo scorso e, cioè, che nella cioè, che nella famiglia dei 27 o 28 Paesi è possibile, anzi è necessario, in alcuni campi, che ci siano livelli di integrazione diversa. Non si può costringere l'Unione europea in tutte le materie a marciare alla velocità del ventottesimo vagone. Se c'è un gruppo di Paesi - in questo caso si tratta di quasi una ventina - che decide, sul terreno della difesa e anche del ruolo geopolitico, di fare un passo più lungo, è positivo che avvenga e naturalmente l'Italia è sempre all'interno di questi formati più avanzati. La terza e ultima decisione di rilievo che viene presa dal Consiglio europeo riguarda il campo della cultura, l'educazione e l'istruzione, rispetto al quale, su spinta del nostro Paese e della Francia, è svolta una discussione, in un recente vertice in Svezia. Da essa sono scaturite alcune decisioni concrete che verranno adottate nel Consiglio europeo, e che riguardano alcune materie che fanno parte di uno di quei motori dell'Unione e della coesione europea, di cui forse discutiamo meno, ma che per l'opinione pubblica, e in particolare per i giù giovani, rappresentano spesso l'essenza stessa dell'Unione europea: la sfida dell'istruzione, la sfida culturale. Le decisioni che prenderà il Consiglio europeo riguardano: in primo luogo, il multilinguismo, con la scelta di uniformare in tutti i Paesi dell'Unione la presenza, oltre alla lingua madre, di almeno due lingue straniere nei diversi corsi di istruzione; decisione non marginale, importante, che offre prospettive anche per la diffusione della nostra lingua, tra l'altro, in diversi Paesi europei. In secondo luogo,

soprattutto per istituzioni culturali e di mobilità. In terzo luogo, concernono la destinazione di fondi molto più significativi al programma Erasmusplus infine, l'individuazione di una rete di università europee, che all'inizio sarà una rete di convergenza tra università europee, più che la costituzione *ex novo* di eccellenze, ma che al suo interno avrà anche il sostegno a università che già oggi svolgono una funzione a livello europeo. Il punto di partenza è che noi abbiamo ottime università nel nostro continente europeo, e ne abbiamo di ottime anche in Italia. Se mettiamo, però, insieme le forze e le competenze, forse possiamo avere livelli di eccellenza in ambito universitario che al momento non sono così immediatamente raggiungibili, e comunque sono raggiunti o da singoli Paesi europei (il Regno Unito) oppure da Stati Uniti, Cina e altri grandi *player* globali. L'Europa può e deve avere un ruolo maggiore da questo punto di vista. Credo che dobbiamo essere orgogliosi del fatto che il nostro Paese su questi temi, come sempre, faccia un po' da apripista, da battistrada e svolga il ruolo di uno di quei Paesi maggiormente convinti che la dimensione dell'Unione europea culturale, dell'istruzione e dell'educazione, sia fondamentale se parliamo dello spirito che deve animare il progetto dell'Unione. Accanto alle decisioni che vi ho appena

partenza di un dibattito - di una discussione sulle prospettive dell'unione monetaria e bancaria europea e su tutti gli aspetti che a questa sono collegati. Sulle politiche migratorie, il punto di partenza - per quanto ci riguarda - è che l'Italia, e non da oggi, si presenta più che mai con le carte in regola e a testa alta alla discussione europea sulla questione migratoria; carte in regola e testa alta che derivano, molto semplicemente, dai risultati che siamo riusciti a ottenere in questo periodo. E questi risultati

Sono risultati talmente evidenti che dovrebbero essere riconosciuti da tutti i Paesi; sostenuti - è il momento di sostenerli - e rivendicati con orgoglio dal nostro Paese. Sono risultati, innanzitutto, sui numeri degli arrivi. Voi sapete che gli arrivi di migranti nel nostro Paese si sono ridotti su base annua del 33 e si sono ridotti negli ultimi cinque mesi, dal primo luglio a oggi, del 69 per cento. Tradotta in termini reali, questa diminuzione dal primo luglio a oggi

lavoro diplomatico; lavoro di costruzione di capacità della Guardia costiera libica; lavoro di rapporti bilaterali con le autorità libiche, lavoro di rapporti con comunità locali, milizie, forze presenti in quel territorio; lavoro ai confini meridionali; lavoro con i Paesi di provenienza o di transito. Dietro queste cifre c'è non una bacchetta magica, ma il lavoro importantissimo svolto dal Governo negli ultimi mesi, che dobbiamo rivendicare

di questo lavoro sul quale oggi stiamo con forza insistendo è quella parte che riguarda le condizioni dei migranti che sono in Libia,

e ottenuto i risultati di cui parlavo, ha avuto tra le sue conseguenze positive che, finalmente, si sono accesi i riflettori sulla situazione dei diritti umani in Libia. È merito nostro. Non è merito di qualcuno che oggi racconta queste cose come se avesse scoperto una realtà imprevedibile! È grazie all'accordo e al trattato tra Italia e Libia che oggi le organizzazioni delle Nazioni Unite sono in grado di essere presenti e di intervenire sul territorio libico.

ha portato i rimpatri volontari assistiti dalla Libia verso altri Paesi africani dalla cifra di poco meno di 3.000 dell'anno scorso alla cifra

A mio parere - ne sono stato testimone diretto sia negli anni scorsi che nelle ultime settimane - c'è stata una straordinaria assunzione di responsabilità da parte di molti Governi africani della situazione. In questo, anche la denuncia delle condizioni umanitarie in Libia ha avuto un impatto positivo, perché ha creato un effetto *shock* nei Governi africani. L'Africa è un continente che fonda la propria identità sul rifiuto dello schiavismo. E, quindi, pensate che cosa possa significare, in un continente come quello, vedere le immagini circolate in questi mesi: ha provocato un cambiamento di atteggiamento. Diversi Paesi, che naturalmente sulle rimesse dei migranti comprensibilmente reggono una parte significativa della propria economia, fanno fatica a raccontare alle loro comunità e alle loro opinioni pubbliche che si fanno dei rimpatri, soprattutto se non sono volontari. E tuttavia, nelle ultime settimane, di nuovo, grazie a quello che siamo stati capaci di iniziare nel rapporto con la Libia e con l'Africa, hanno aperto la strada - lo si è visto al vertice di Abidjan

La domanda che quindi rivolgeremo ai nostri amici dell'Unione europea, nel corso della discussione che si farà sui temi migratori, è se su questi risultati - lo dico con orgoglio, ma anche aggiungendo la parola purtroppo - che sono prevalentemente risultati dell'azione italiana, sia pure sostenuta economicamente dalla Commissione europea, dalla Germania e da qualche altro Paese, ma non certo dall'insieme degli Stati membri, neanche sul terreno economico,

giusto per citare un dato - che il gruppo dei quattro Paesi di Visegrád (Ungheria, Cechia, Slovacchia e Polonia), che è quello più distante da noi, se parliamo della dimensione interna delle migrazioni,

se ognuno, in proporzione al proprio bilancio, desse una cifra di questo genere, saremmo in grado di accompagnare l'azione dell'Italia con le risorse necessarie, e sarebbero in questo caso sufficienti. Questo gruppo di Paesi ha deciso di accompagnare l'azione italiana nella dimensione esterna con questo stanziamento io non ho alcuna remora a dire che lo considero un fatto positivo. Questo non cambia in nulla la nostra posizione politico-culturale, non apre alcun varco all'idea che si possa abbandonare quel principio di obbligatorietà della solidarietà nei confronti dei rifugiati che l'Unione europea ha dichiarato e non è mai riuscita ad attuare. La posizione italiana non cambia di una virgola da questo punto di vista, deve essere molto chiaro. Al tempo stesso, però, se si allarga la disponibilità a riconoscere l'importanza di quello che stiamo facendo sulla dimensione esterna, credo sia molto importante. Andiamo quindi a questa discussione, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, con l'orgoglio di essere contemporaneamente il Paese che dà il buon esempio in Europa nell'ambito della

come quello migratorio, centrale nella discussione europea del 2018: il tema del futuro dell'Unione monetaria, dell'Unione bancaria e delle prospettive che si aprono da questo punto di vista.

nella seconda metà di giugno del 2018 - uso il condizionale perché sono già sul tappeto delle spinte e delle tendenze a prendersi un tempo più lungo, ma vedremo ma vedremo - comincia innanzitutto sulla base di proposte della Commissione. La Commissione ha fatto un pacchetto di proposte che l'Italia considera - come ho detto anche al presidente Juncker, apprezzando lo sforzo e l'impegno della Commissione da questo punto di vista - come una buona base di partenza. Tradotto dal gergo diplomatico, dire «buona base di partenza» vuol dire che noi apprezziamo lo sforzo fatto dalla Commissione e consideriamo che i temi che quelle proposte affrontano sono quelli che è giusto oggi mettere in discussione. Riteniamo anche che su queste medesime proposte si possa e si debba andare più avanti, consapevoli - onorevoli senatrici e senatori - che un pezzo rilevante della famiglia europea vorrebbe andare più indietro, non più avanti, rispetto ad esse. Già nelle discussioni preparatorie del del Consiglio europeo c'è stata una discussione piuttosto evidente tra posizioni che potremmo chiamare centro-nordiche e posizioni che potremmo chiamare mediterranee, con accenti diversi - per semplificare

È decisivo che si crei un meccanismo di riserva - in gergo si dice un meccanismo di *backstop* - dell'unione bancaria, che sia comunitario comunitario e non affidato alle decisioni di singoli Stati. Il che vuol dire - cosa di cui non abbiamo potuto servirci nei mesi scorsi - che, di fronte a delle crisi bancarie che coinvolgono questo o quel Paese, c'è un meccanismo comunitario di riserva che copre ampiamente siffatta possibilità. è l'idea di un Ministro delle finanze europeo, ma a condizione naturalmente che

trasformarsi in una specie di controllore della contabilità di economie di questo o quel Paese e preferibilmente dei Paesi dell'Europa mediterranea o meridionale. Questa seconda cosa ci farebbe dire: «no, grazie». Si dovrebbe accompagnare finalmente a una politica di bilancio comune, una politica che finalmente può anche avere delle risorse proprie a disposizione. E su questo ci ha lavorato molto una commissione presieduta dal senatore Monti, alcuni anni fa.

di investire sui beni pubblici, sui beni comuni - ognuno li chiami come preferisce - europei. Noi abbiamo bisogno di avere capitoli di bilancio comuni europei che ci consentano di affrontare temi come le migrazioni, la sicurezza la difesa, e mettano in piedi meccanismi di assicurazione sociale. L'Italia - per esempio - ha proposto un meccanismo di assicurazione sociale contro gli *shock* asimmetrici sul terreno dell'occupazione, e cioè quando in un Paese a causa di una crisi si crea un problema occupazionale specifico. Che bello Che bello sarebbe uno strumento di questo genere, finanziato da risorse proprie dell'Unione europea. Sarebbe un contributo fondamentale alla convergenza. Avviandomi l'obiettivo è sul tappeto, i temi sono sul tappeto. Si tratta di cogliere l'occasione costituita molto semplicemente dal fatto che, dopo una crisi economica molto rilevante, l'Unione europea, e l'eurozona in particolare, attraversa un periodo di crescita stabile e diffusa in tutti i Paesi. Ieri l'OCSE ha addirittura affermato che questa crescita è particolarmente accelerata in due Paesi: il primo è la Germania e il secondo

suscitare discussioni inutili: noi siamo ancora al di sotto della media europea di crescita nel 2017. Il rapporto dell'OCSE parla di velocità, di ritmo di questa crescita. Ma questo ritmo e questa velocità sono un fatto incoraggiante per le nostre imprese e potenzialmente incoraggiante, se lavoriamo bene per la società, per il lavoro, per i problemi sociali che abbiamo davanti.

favorevole per qualche ulteriore misura di natura contabile che, al limite, rischia di provocare delle crisi, invece che sanarle e prevenirle? Certamente no. Il punto è se abbiamo la forza e la capacità di usare questa situazione favorevole per proseguire nella strada che abbiamo seguito in questi anni di rispetto delle regole fissate dall'Unione, e per spingere l'Unione a una politica più espansiva, di maggiori investimenti, di maggiore autonomia del proprio bilancio, di maggiore capacità di una politica migratoria comune, di convergenza.

per la semplice ragione che non correggere gli squilibri macroeconomici dei Paesi in *surplus* danneggia l'intera economia europea e a lungo andare anche quei stessi perché investire servirebbe ai Paesi in *surplus* al loro interno, oltre che a dare ossigeno ai mercati e agli investimenti su scala europea. l'Italia fa parte di questa stagione tutto sommato positiva dal punto di vista macroeconomico; poi conosciamo le difficoltà che abbiamo sul piano sociale, i problemi che dobbiamo affrontare e risolvere, lungi da me metterli in secondo piano.

E faremo di tutto anche nel prossimo Consiglio europeo per spingere l'insieme dell'Unione a cogliere questa occasione in positivo per lo sviluppo e per il lavoro.

e vorrei mettere in luce due conseguenze per l'Italia derivanti dalla situazione a livello europeo che lei ha descritto in modo, a mio avviso, persuasivo. Il primo punto è l'atteggiamento dell'Italia nei confronti dell'Unione europea. tra noi più favorevoli all'Unione europea e che vorrebbero più Europa possono trarre incoraggiamento dall'evoluzione - che lei a grandi linee ha descritto - avvenuta negli ultimi diciotto mesi dopo il voto su Brexit. Non c'è stata diffusione degli atteggiamenti divorzisti - come lei li ha chiamati - e c'è stata un'unità tra i 27, nel negoziato con il Regno Unito, molto maggiore di quella che ci si poteva aspettare. Va sottolineato però che non sono ancora consolidati i motivi di sollievo che, in diverse tappe, nel corso di questi ci hanno portati a ritenere che la situazione dell'Unione europea si stesse rafforzando. Questo, in parte perché i migliori atteggiamenti sono dovuti - come lei ha messo in luce - alla congiuntura economica più favorevole, perché - non dimentichiamolo - a ogni elezione nazionale stiamo con l'orecchio teso e l'occhio attento per vedere cosa fanno i partiti meno favorevoli all'Unione europea e non è che sia una serie ininterrotta di trionfi per gli europeisti.

secondo me, dovrebbero riflettere, perché il decorso dell'Europa negli ultimi diciotto mesi, in particolare dopo Brexit, mette in luce insegnamenti molto importanti sull'Italia. Perché? Perché? Molte volte abbiamo sentito dire - credo in assoluta buona fede - che bisogna andare a Bruxelles con un altro *animus*: negoziare diversamente, battere i pugni sul tavolo, tenere sempre presente e far valere la minaccia che il nostro Paese potrebbe uscire dell'Unione europea. Abbiamo assistito all'esperienza Brexit, quella di un Paese che ha deciso, con modalità democratiche, di uscire dall'Unione europea. È il Paese, con tutto il rispetto per il nostro e per altri, più dotato storicamente di grande capacità e abilità di negoziato, di grandissima forza d'urto, se mette insieme il proprio potere economico, diplomatico e politico; eppure abbiamo visto come un atteggiamento inizialmente spavaldo e di durezza si è risolto, da molti punti di vista, in uno scioglimento della posizione dell'Unione europea. Proviamo a immaginarci, cari colleghi meno di me e meno di noi favorevoli e sensibili all'Unione europea, che cosa avverrebbe all'Italia, a un Governo italiano, se per caso fossero prese seriamente come sempre bisogna sul piano dell'onestà intellettuale - le proposte di chi dice "andiamo a sbattere i pugni sul tavolo" o "al limite minacciamo l'uscita dall'Unione europea". Abbiamo avuto la fortuna di avere in questi diciotto mesi un *test* di laboratorio di cosa avverrebbe di fronte a tali atteggiamenti. La seconda e più breve considerazione, signor Presidente del Consiglio, riguarda l'avvio delle discussioni sulla riforma dell'Unione monetaria, In particolare ha espresso un dilemma che ho trovato molto interessante quando ha detto: a cosa deve puntare l'Italia? Ad avere qualche misura contabile in più, che al limite può far peggiorare la situazione del Paese? Oppure abbiamo la forza e la capacità di sfruttare questa stagione, tutto sommato positiva (sono parole sue), per dare un contributo alla riforma della zona euro buono per l'Europa e buono per l'Italia? Mi sembra che lei non abbia dubbi nel puntare sulla seconda direzione. Pertanto, vorrei dirle che in un momento in cui la Commissione fa proposte generose e articolate come quella del Ministro delle finanze per l'eurozona, credo non si possa perdere questa rarissima occasione per far valere - finalmente - la logica economica e politica che sta a cuore all'Italia, quella cioè - lei l'ha ripetuto più volte - di dare una dignità di trattamento agli investimenti pubblici seri, monitorati e verificati come tali.

(poi ognuno ha il suo giudizio sull'uso che è stato fatto di questa flessibilità) - vi diciamo: non è questa la strada, la scorciatoia su cui l'Italia vuole procedere anni. Vi chiediamo di inserire stabilmente gli investimenti pubblici tra le legittimità del Patto di stabilità e proponiamo che in futuro tutti si rinunci a una flessibilità lo abbiamo visto - si trasforma, per l'inevitabile pressione politica che esiste in ogni Paese, in più *bonus* e trasferimenti e meno investimenti pubblici. Credo che questo sia un contributo

spero anch'io, come è stato da lei suggerito, che giovedì e venerdì il vertice europeo possa essere un punto di riferimento obbligato e soddisfacente. Rievocando però il percorso della Brexit, mi pare che si sia da lei accennato, con immagine letterariamente brillante, a un duplice *shock* incassato dall'Europa: quello della Brexit e quello dell'elezione di Donald Trump. Ovviamente, immagino che lo tra virgolette perché quando votano grandi democrazie, come sono entrambi i Paesi, nessun risultato può essere scioccante. A proposito del rapporto con Trump, mi ha un po' sconcertato ascoltare da lei, oggi,

un gesto di grande miopia e scarsa responsabilità. A questo proposito, uso una sua immagine: l'Unione europea non deve essere costretta a marciare alla velocità del ventottesimo vagone. È giusto, ma è anche vera

Non ci nascondiamo dietro le colorate e colorite iniziative del presidente Trump. La linea politica italiana ed europea è stata, negli ultimi dieci anni, su questo grande problema, a nostro giudizio, del tutto sbagliata. Lei considera uno *shock* - e forse ha ragione - che Trump abbia vinto la sfida con la Clinton; ma lei deve anche rispettare quegli italiani e quegli europei che hanno considerato altrettanto scioccante per otto anni, quando si apriva la sezione delle Nazioni Unite, ascoltare la delegazione americana avere come priorità il diritto al nucleare e il connesso diritto all'antisemitismo da parte di Teheran. Né in questi otto anni abbiamo ascoltato adeguate prese di posizione europee di tutt'altro senso. Mi permetto, ripassare gli appuntamenti di giovedì e di venerdì: una rete di università europee. Signor Presidente del Consiglio, non abbiamo nulla in contrario, siamo favorevolissimi; ma ci vergogneremmo se in questa rete di università europee fossero comprese quelle che, con il compiacimento della vice presidente Mogherini, nei mesi scorsi, hanno compiuto atti di quello che loro chiamano antisionismo (ma i confini con l'antisemitismo sono molto sfumati) nei confronti di prestigiosi docenti e ricercatori di università israeliane. Veniamo all'altro punto: i migranti. Noi siamo all'opposizione, ma condividiamo tutte le sue parole sull'orgoglio dell'Italia per aver visto ridursi di 80.000 unità questo flusso. Abbiamo anche un certo orgoglio nel constatare come nella comunità internazionale non siano mancati apprezzamenti

credere a scatola chiusa, ma su cui il Governo ha il diritto e il dovere di fare chiarezza. Si rimprovera all'Italia un eccesso di fiducia nell'unità nazionale libica; si attribuisce all'Italia un patto di omertà con la Guardia costiera libica; si attribuisce all'Italia una certa complicità in questo orientamento, degno della peggiore UNESCO, nell'aver trasformato questi campi libici in campi di autentica tortura. Per questo, augurando all'Italia di esprimere il proprio punto di vista, con grande dignità, al prossimo vertice di giovedì e venerdì, noi riteniamo che questo non sia per l'Europa un momento particolarmente brillante. Se è consentita una considerazione cronistica, mi chiedo perché la Mogherini non ha pronunciato neanche una frase sull'attentato a New York. Perché tanto compiacimento con questa pace palestinese, che ormai - lo sappiamo tutti - significa con Hamas? Perché si è dimenticata - e vuole che l'Europa dimentichi - che tanto Hamas quanto Hezbollah

alla quale - glielo ricordiamo come Gruppo Lega tutte le volte che viene in Senato - il suo predecessore non ci aveva abituati. La ringrazio molto per il rispetto che dimostra nei confronti del Senato della Repubblica

che, nel momento in cui si è parlato di difesa europea, di Forze armate europee e di difendere o comunque tutelare i confini dell'Europa,

potrebbe essere alla vostra attenzione nei prossimi giorni la decisione degli Stati Uniti di spostare la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Abbiamo visto un'alzata di scudi a livello internazionale, anche da parte di alcuni Stati europei, e delle dichiarazioni di ostilità nei confronti degli Stati Uniti per questa decisione. Noi siamo dell'idea che Israele debba essere lasciato libero di decidere sul proprio territorio nazionale la propria politica interna e, in particolare, quella estera. Di conseguenza, nel momento in cui gli Stati Uniti, insieme ad Israele, decidono che l'ambasciata statunitense venga venga spostata a Gerusalemme, devono essere lasciati liberi nella gestione di questa decisione.

debba scoraggiare l'uso della forza nel caso di rivendicazioni di autonomia o di indipendenza. L'Europa e gli Stati europei devono diventare un interlocutore importante e affidabile,

Per quanto riguarda poi il discorso della cultura, dell'educazione e delle questioni sociali, siamo sicuramente dalla sua parte quando ci parla di implementazione del programma Erasmus, quando ci parla di università europee e, di conseguenza, la appoggiamo in questa *mission* appoggiamo in questa *mission* che vuole portare avanti. Siamo anche dell'idea che debbano essere estesi i diritti negli Stati membri dell'Europa, ma in questa estensione riteniamo che debba essere lasciata autonomia agli Stati membri. Siamo dell'idea che debba debba essere presa in considerazione la risoluzione dei diritti dei bambini del 21 novembre scorso presso le Nazioni Unite, una risoluzione importante cui è stato dato poco risalto. Chiediamo di farsi portavoce in Europa di questa risoluzione.

ci lascia perplessi e ci spaventa, visto che abbiamo notato che dalla Tunisia non arrivano delle personcine proprio affidabili. Molto spesso dalla Tunisia arrivano *ex* galeotti e persone che non vengono nel nostro Paese con i fiorellini in mano. in mano. Presidente, riteniamo debbano essere coinvolti maggiormente i Paesi rivieraschi sul Mediterraneo, ma anche quelli di partenza come il Niger, dove sono state fatte delle politiche di cooperazione internazionale molto importanti e che, in alcuni casi, hanno avuto successo.

equità. I soldi che spendiamo per tenere negli alberghi queste persone potrebbero essere utilizzati meglio per poter accogliere in maniera più adeguata chi scappa da una guerra, chi realmente ha diritto a stare nel nostro Paese e che noi abbiamo il dovere e la volontà di accogliere.

Questo accordo deve essere modificato e non possiamo pensare che tutti vengano portati nel nostro Paese perché non possiamo pensare che tutto sia sulle nostre spalle. Presidente, c'è un'altra cosa che ci lascia perplessi e anche questo, secondo noi, deve essere portato all'ordine del giorno e deve essere portato all'attenzione di chi ci ascolta in Europa. Molti dei migranti, spesso finti profughi, anziché essere riconoscenti a chi li accoglie, spacciano droga e violentano le nostre donne e vengono nel nostro Paese a fare ciò che vogliono. Non possiamo pensare che, quando vengono presi e condannati, non vengano rimpatriati. Presidente, rimpatriate almeno

Presidente, per quanto riguarda i rimpatri, ricordo che state rimpatriando 5.000 persone all'anno, su 700.000 che sono entrate nel nostro Paese. Il ministro Maroni, a suo tempo, ne rimpatriava molte di più, con un decimo degli arrivi nel nostro Paese. *(Applausi dal un po' più d'impegno per essere credibili in Europa. Infine, ho visto che lei ha esaltato la crescita del nostro Paese. Ha perfettamente ragione, d'altronde stanno crescendo tutti, tutta l'Europa sta crescendo. Il problema

progressi compiuti negli argomenti posti al centro della cosiddetta «agenda dei *leader*», elaborata dal presidente Donald Tusk, Tusk, ed approvata dallo stesso Consiglio in data 27 ottobre 2017, cui hanno fatto seguito una serie di incontri bilaterali tra lo stesso presidente

si tratta del secondo *summit* per discutere di difesa, assetti sociali e culturali dell'Europa, migrazione e, infine, di Europa economica e monetaria, nonché di unione bancaria. Argomento, quest'ultimo, che è tuttavia subordinato, secondo gli accordi presi, alla realizzazione dei nuovi assetti istituzionali che dovrebbero nascere nell'Eurozona: bilancio europeo, Fondo monetario europeo, istituzione di un Ministero del tesoro europeo ed infine inserimento del *fiscal compact*

per quanto riguarda lo *status* dei cittadini europei residenti nel territorio inglese ed il contenzioso finanziario relativo ai debiti pregressi della Gran Bretagna, mentre rimane sullo sfondo il tema dei rapporti con Dublino e la ricaduta delle eventuali decisioni sullo *status* della Scozia e della City. Per quanto riguarda i problemi della difesa è necessario avviare quanto prima un sistema comune che faccia fronte alle difficoltà che si intravedono nei rapporti con gli Stati Uniti, sia per quanto riguarda la NATO, ma soprattutto le più recenti divergenze a proposito della politica mediorientale, dopo la decisione del presidente Donald Trump di spostare la sede dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. Decisione che comporta, di fatto, il riconoscimento di Gerusalemme come capitale esclusiva dello Stato d'Israele, in aperta contraddizione con le tesi europee secondo le quali Gerusalemme deve continuare ad essere la capitale dei due Stati: Israele Sugli aspetti legati alla politica sociale è necessario prendere atto delle divergenze che si sono prodotte tra i diversi Paesi membri, al fine di individuare quelle politiche che mirano ad un loro superamento. Essendo diverse le posizioni di partenza, non è pertanto possibile individuare una politica una politica univoca, che non tenga conto delle sottostanti diversità. Secondo le stesse valutazioni della Commissione europea vi sono Paesi come la Germania, l'Olanda o Malta che hanno un tasso di disoccupazione inferiore o prossimo al 4 che gli economisti indicano al di sotto del limite frizionale, mentre altri, come la Grecia, la Spagna che superano o sono prossimi al 20 per cento, ed altri ancora come l'Italia, la Francia, il Portogallo o Cipro che superano o sono prossimi al 10 per cento. Occorrerà, pertanto, analizzare le cause che le cause che determinano queste diversità di valori: se esse sono legate a fatti strutturali (come sembra essere evidente in Grecia), alla scarsa competitività macroeconomica (come nel caso della Francia) oppure alle cattive politiche congiunturali, come in Italia, imposte da un eccesso di *austerity* che non consente il pieno utilizzo dei fattori produttivi, come risulta evidente dal *surplus* delle delle partite correnti della bilancia dei pagamenti. Sul problema delle migrazioni non si può non prendere atto delle parole di Juncker, secondo il quale nel Mediterraneo l'Italia ha salvato l'onore dell'Europa. Riconoscimento giusto e gradito, al quale, tuttavia, devono seguire fatti concreti sia per quanto riguarda la distribuzione dei richiedenti asilo sia circa lo sviluppo di una politica europea a favore delle zone d'emigrazione - soprattutto in Africa - al fine di rimuovere le condizioni sociali che determinano un esodo così drammatico e doloroso. È necessario che l'Europa investa in questi Paesi,

Il punto che per l'Italia riveste, comunque, maggiore importanza è il futuro dell'Eurozona, specie dopo le ultime prese di posizione del presidente della Commissione Juncker. Nessuna obiezione sulla necessità di un rafforzamento delle istituzioni Questa prospettiva costituisce, al contrario, l'unico strumento per arrestare il suo più recente declino e colmare il fossato che si è aperto con vasti strati dell'opinione pubblica, molti dei quali hanno smarrito il senso stesso dello stare insieme. Il tema è "quale istituzione", per "quale politica", signor Presidente. Se non si chiarisce questo legame, la riforma, pur necessaria, scade nella semplice ingegneria costituzionale, che non solo rischia di non ottenere alcun risultato, ma di produrre contraddizioni ancora maggiori. Va bene, quindi, un diverso bilancio, seppur nella formula riduttiva indicata da Juncker, come va bene il Fondo monetario europeo, in sostituzione dell'ESM, il Fondo salva Stati, a condizione tuttavia che non si pensi a una struttura tecnocratica che esautori i poteri della Commissione nella valutazione, a tutto campo, delle politiche economiche dei Paesi membri. Al tempo stesso, nessuna contrarietà a un Ministro del tesoro che sappia cogliere la complessità della situazione europea e individuare quelle politiche indispensabili per rimettere in il *fiscal compact* nell'ordinamento europeo, occorre discutere con grande determinazione, signor Presidente. L'articolo 16 del Trattato istitutivo, firmato da tutti i Paesi con la sola eccezione della Gran Bretagna e della Repubblica Ceca, prevedeva che dopo cinque anni, quindi nel 2018, si procedesse a una valutazione dell'esperienza maturata, prima di procedere oltre sulla strada del suo inserimento nell'ordinamento comunitario. Questa fase non può essere bypassata. Vi sono ovvie ragioni di carattere giuridico: le regole vanno sempre rispettate, specie se hanno la veste particolarmente solenne di un trattato internazionale; ma sono quelle economiche che impongono ancor di più una simile verifica, anche se la Commissione europea non sembra volersi attivare. Sarebbe stato, infatti, opportuno avere a disposizione una sua valutazione sui successi (pochi, invero) conseguiti e le contraddizioni (molteplici) che si sono manifestate. Recentemente un bilancio è stato tentato da alcuni economisti della BCE. Secondo questo studio, i *fiscal criteria*, previsti dalle regole del *fiscal compact*, sarebbe stati rispettati solo da cinque dei 29 Paesi, a dimostrazione di quanto possano essere astratte determinate formulazioni che considerano alcuni aspetti della politica economica come vere e proprie variabili indipendenti, ossia del tutto avulse da un più generale contesto macroeconomico. tratta di un errore di metodo che porta, inevitabilmente, al mancato rispetto delle regole stesse. È necessario pertanto, signor Presidente, capire Non si tratta, infatti, di respingere le regole in quanto tali. La solidità finanziaria è un requisito indispensabile ai fini del contenimento del debito pubblico, ma lo è anche la crescita del denominatore, vale a dire il PIL nominale sulla cui base si calcola il relativo rapporto. Se il tasso di crescita reale è troppo basso, se la deflazione se la deflazione dei prezzi prende il posto dell'inflazione, quel rapporto non è destinato a diminuire, ma a crescere, nonostante le politiche di austerità messe in atto. È allora indispensabile trovare quel giusto equilibrio tra gli andamenti di finanza pubblica e quelli e quelli dell'economia reale per giungere al *mix* più opportuno per ottenere, al tempo stesso, più benessere e il progressivo risanamento finanziario, specie per quei Paesi che presentano un attivo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti: sintomo vistoso di una sottoutilizzazione dei fattori produttivi esistenti al loro interno, a partire dal lavoro. L'esperienza empirica dimostra che una regola uniforme non può valere per tutti i sistemi economici e per tutte le fasi della congiuntura. La Francia,

correnti della bilancia dei pagamenti. La Spagna, a sua volta, è stata in procedura d'infrazione dal 2009. L'Italia si trova, invece, in una situazione opposta. Ha sempre rispettato, seppure con qualche fatica,

debito-PIL, che non accenna a diminuire, ma con un attivo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti che è un multiplo del suo tasso di crescita. il Governo deve quindi operare in una direzione coerente con le premesse enunciate, facendo valere le buone ragioni di un Paese, come l'Italia, che in tutti questi anni ha dimostrato, a differenza di altri, il suo rispetto per le regole, per quanto non condivise; sollecitando l'unione bancaria a fare il possibile per superare manovre dilatorie da qualunque parte provengano, al fine di ridare fiducia ai risparmiatori ed evitare che la relativa "incompiuta" - soprattutto la mancata garanzia europea per i depositanti possa alimentare nell'opinione pubblica il sospetto che l'Europa non sia una struttura realmente democratica, ma solo un grande mercato dominato dalla legge del più forte. Comunque, signor Presidente,

Ebbene, siamo alla conclusione della legislatura e, quindi, dal mio punto di vista l'occasione è propizia per una sorta di promemoria, a partire da quella che a me sembra una premessa di ordine metodologico necessaria, alla quale seguiranno alcune osservazioni su taluni nuclei tematici a nostre avviso fondamentali. Il Consiglio europeo si riunisce in via ordinaria quattro volte all'anno. Il Trattato stabilisce che il Presidente del Consiglio assicuri la preparazione e la continuità dei lavori, in cooperazione con il Presidente della Commissione

Quindi, io mi domando, sotto il profilo delle modalità di procedimento, che senso abbia, alla vigilia e nell'imminenza del Consiglio europeo, definire orientamenti e indicazioni che andrebbero meglio approvati in un momento precedente, quando, in qualche misura, sia ancora possibile vincolare e indirizzare le scelte del Governo in ambito europeo. Questo non è un appunto riservato direttamente a lei, signor Presidente, ma è una considerazione di carattere più generale. Noi abbiamo ascoltato con la dovuta attenzione le sue argomentazioni. Lei ha il pregio di saper argomentare, che non è poco. pare, però, che non abbia sufficientemente accentrato la sua attenzione in ordine a tre antefatti che mi paiono assolutamente significativi in questa temperie politica e di relazioni internazionali: innanzitutto, la scelta del presidente Trump di riconoscere Gerusalemme, che il diritto internazionale considera una città condivisa, nella parte Ovest israeliana ed Est palestinese, come la capitale del solo Stato d'Israele, un atto che a nostro avviso risulta irresponsabile e foriero di gravissimi pericoli per la pace, un atto che non è in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, che non aiuta - per usare un eufemismo - una prospettiva di pace della regione, che rischia di alimentare tensioni, contrasti, contrapposizioni, persino di dare fiato a nuove stagioni, ahimè, di impronta terroristica. Peraltro, è una posizione costante dell'Unione europea che Gerusalemme deve essere la capitale sia dello Stato d'Israele che di quello palestinese, quindi un impegno da parte dell'Europa e da parte nostra per favorire questo processo di *State building* palestinese. Il secondo antefatto sul quale lei secondo me ha sorvolato si è svolto il 29 e 30 novembre ad Abidjan: alludo al *summit* tra l'Unione europea e l'Unione africana, perché se è vero che la questione africana sarà la grande, centrale questione del XXI secolo, è evidente che questo dato interroga sia il nostro Paese, sia l'Unione europea perché ci sia un impegno corposo di investimenti in vista della creazione di opportunità economiche e occasioni di lavoro nel continente africano. Ebbene, nel corso di questo vertice, è stato messo in luce anche il trattamento dei migranti africani che in molteplici casi - ma su questo tornerò vengono imprigionati, torturati, se sono donne stuprate da parte di trafficanti di esseri umani e spesso venduti come schiavi. C'è un terzo aspetto: la questione della Brexit e l'accordo che è stato raggiunto l'8 dicembre, sul quale tornerò in conclusione. Ho detto che accentrerò due o tre *focus* su questioni a mio avviso centrali. La prima è il tema delle proposte in campo di politica economica e finanziaria, la cui bussola di orientamento non può che essere il tema della ripresa e della crescita. A me pare che sia necessaria una correzione, un ripensamento, una rinnovata declinazione del tema del *fiscal compact* e l'avvio di una riscrittura che vada nella direzione di una *golden rule* relativa a spese d'investimento e soprattutto a spese che consentano il decollo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. Se è vero - recentemente ho presentato, con Valerio Castronovo, un libro sulla politica estera tedesca - che siamo tutti per una Germania europea e non per un'Europa tedesca, il tema, ad esempio, della riduzione almeno al 3 per cento del limite massimo per il saldo di bilancia commerciale di ciascun Paese membro e l'introduzione di sanzioni corrispondenti a quelle previste per *deficit* di bilancio eccessivi, è un tema a mio avviso assolutamente fondamentale se si vuole puntare ad un riequilibrio dei ruoli e dei protagonismi. Il tema della ripresa e della crescita non può essere estraneo alla proposta della emissione di titoli di debito europeo garantiti da tutti gli Stati membri alla necessità di definire un piano per l'Eurozona di investimenti pubblici che abbiano un alto significato sociale e di riqualificazione e ripristino del territorio, delle periferie urbane, dei luoghi della fragilità e della

Potrei continuare, ma è il tema dell'immigrazione quello sul quale, a mio avviso, la sua esposizione ha peccato di un eccesso di ottimismo e di un limite di realismo. È recente l'audizione in Commissione affari esteri di due incontri con esponenti dell'UNHCR e dell'Organizzazione internazionale per Oggi abbiamo saputo della conferenza stampa di Amnesty International a Bruxelles, che definisce e raffigura un quadro molto più doloroso e molto più problematico di quello che ci è stato descritto. A titolo di esempio, potrei dell'apertura immediata di corridoi umanitari di accesso in Europa, per consentire canali di accesso legali e controllati attraverso i Paesi di transito ai rifugiati che fuggono da persecuzioni, guerra e conflitti, l'impegno a mettere fine alle stragi in mare, le responsabilità della guardia costiera libica, come è emerso da un filmato che riguarda la tragedia consumata il 6 novembre, dove viene plasticamente raffigurato il naufragio dell'Europa e di una civiltà umana consapevole delle proprie responsabilità. l'implementazione rapida del programma di ricollocamento in realtà non ci consegna un bilancio di valutazioni positive; la necessità di affiancarlo alla creazione di adeguate strutture per l'accoglienza e l'assistenza. Vanno poi previste adeguate sanzioni nei confronti dei Paesi come l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica ceca, che non rispettano i vincoli europei. Certamente noi abbiamo avuto un ruolo significativo in Libia. Sotto questo profilo non posso negare la veridicità di alcune sue osservazioni, ma fino a quando non sarà garantito il pieno rispetto della dignità e dei diritti, è evidente che gli accordi con quei Paesi debbono essere ridiscussi, condizionati e, nel caso estremo, sospesi. Il Consiglio europeo metterà sul tappeto i grandi temi della politica estera. Mi ha stupito non sentire un riferimento alla Turchia e al ruolo che l'Unione europea deve assumere nei confronti della Turchia affinché sia posta fine alla repressione contro le opposizioni democratiche, la magistratura, la stampa e le minoranze presenti nel Paese. Vedo che il tempo è tiranno, quindi mi limito a una sola battuta conclusiva senza addentrarmi nei temi molto intriganti e impegnativi della politica comune di difesa europea e della politica di sviluppo della cultura e della ricerca. alla questione della Brexit. Non c'è dubbio che l'accordo cui ho fatto riferimento segni un passaggio significativo, ma bisognerà soprattutto guardare alla condizione dei cittadini italiani in modo che sia assicurata la tutela dei loro diritti. Sono 600.000 i cittadini italiani che risiedono nel Regno Unito e 3 milioni i cittadini

abbiamo ascoltato con grande attenzione le sue comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. Abbiamo ascoltato tante cose, tutte importanti, su un ordine del giorno certamente significativo: il tema della cooperazione strutturata e permanente della difesa europea, le conclusioni del vertice di Göteborg, le politiche inerenti alle migrazioni; temi di cui abbiamo parlato anche l'ottobre scorso, in vista del precedente vertice. Certamente, il Consiglio europeo a proposito di politica estera, non potrà esimersi dal discutere sul fatto nuovo avvenuto pochi giorni fa: mi riferisco alla dichiarazione del presidente Trump di riconoscere unilateralmente Gerusalemme quale capitate esclusiva dello Stato di Israele. Sappiamo quanto questa dichiarazione non sia conforme alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Non promuove la prospettiva di pace in quelle latitudini e apre lo scenario di uno scontro diplomatico in seno all'ONU e l'inizio di un braccio di ferro che potrebbe durare anche a lungo. La crisi di Gerusalemme interroga anche l'Europa che, a conclusione della visita in Europa del *premier* ebraico Netanyahu, registra una presa di distanza da quella decisione, affermando che nessun Paese dell'Unione europea seguirà la decisione degli Stati Uniti su Gerusalemme, compresa l'idea di trasferire la sede dell'ambasciata a Gerusalemme. tuttavia, incendia il Medio Oriente, già fortemente instabile, e trova anche nelle dichiarazioni del presidente russo Putin, il quale ad Ankara ha approvato la campagna antiamericana del presidente turco Erdogan, motivi di preoccupazione. A cascata è intervenuta la Lega araba, il Marocco minaccia una mobilitazione mondiale il 23 dicembre, la Giordania - sempre amica - non dà a Israele il permesso di riaprire l'ambasciata ad Amman, ufficialmente con la scusa di problemi d'ordine pubblico. Non sappiamo, al momento, quali siano le reazioni di egiziani e sauditi, ma perfino parte della Destra israeliana è preoccupata non del "se", perché è un regalo quasi insperato, ma del "quando". Con l'Iran alle soglie, il Libano instabile, i palestinesi riunificati, il Sinai sotto scacco ISIS, ci si interroga se fosse proprio questo il momento per dare seguito a una promessa elettorale. Anche se è ancora troppo presto per fare bilanci, la situazione resta delicata e il rischio è che il minimo incidente possa innescare ulteriori terribili violenze. Hamas ha chiamato a una nuova *intifada* e, anche se i palestinesi sembrano fiaccati dal subire un impoverimento costante, sia economico che sociale, e quindi poco reattivi a mettere in piedi una terza *intifada*, gli scontri che si sono avuti fino a oggi tra israeliani e palestinesi ci devono trovare attenti e sensibili a quanto succede attorno a noi per poter essere catalizzatori e costruttori di pace, e costruttori di pace, mettendo l'Unione europea nelle condizioni di discernere, di ragionare, di non sposare le mode, ma di saper condannare equamente e di confermare in confini sicuri lo Stato di Israele. Ecco, il tema della cooperazione strutturata delle politiche estere europee si pone con sempre maggior urgenza. Trovo interessante, signor Presidente, quanto riferito a proposito del vertice di Göteborg. Qui la costruzione europea ha ripreso i principi fondamentali, rendendo omaggio ai padri fondatori dell'Europa Schuman, De Gasperi, Adenauer. Gli studenti d'Europa, gli universitari d'Europa, i ricercatori d'Eropa, i docenti d'Europa: siamo d'accordo. Sentire che il vertice abbia sancito il principio che le persone stanno al primo posto mi sembra una bella affermazione di umanesimo, del tutto necessaria in un tempo, come quello odierno, dominato dal primato della finanza e della tecnica fredda e spersonalizzata. spersonalizzata. Mi consenta però, a proposito di università: come si fa a parlare di atenei europei e quindi di sistema europeo degli atenei, se i nostri ragazzi sono ancora obbligati all'iscrizione a molti corsi di laurea a numero chiuso, favorendo così l'emigrazione dei nostri studenti verso altri Paesi, che sono felici di accoglierli, per l'incidenza che lo studentato produce sul prodotto interno lordo nazionale di quei Paesi dal punto di vista culturale ed economico? Speriamo che l'università europea non voglia dire solo altri costi a spese del nostro sistema d'istruzione, dei nostri ricercatori e docenti precari. Non si può non essere d'accordo quindi con l'approvazione del Pilastro sociale europeo. Era ora che il linguaggio europeo declinasse in una carta fondamentale principi fondamentali e diritti in tema di pari opportunità e condizioni di lavoro eque (protezione, inclusione sociale, pensioni, uguaglianza di genere). È bello apprendere che finalmente l'Europa si convinca che la forte protezione sociale per le persone può procedere di pari passo con la competitività economica. Per cui quando il presidente Juncker afferma che è il momento di far nascere un'Europa sociale ed è ora di mettere le persone al primo posto, noi non possiamo non essere d'accordo. Tutto questo però non può e non deve restare un'affermazione inscritta all'interno di una Carta, seppure con la dignità di una Carta fondamentale, ma deve tradursi in rispetto preciso per quelle che saranno le elaborazioni dei singoli Paesi riguardo la centralità della persona in tutte le azioni

dei nostri posti di lavoro, ci si aspetta che l'Unione non gridi allo scandalo, ma riconosca che dietro ad ogni azione di questo tipo c'è la difesa della persona nel suo essere integrale, destinatario di sostegno e tutela concreti e, non di un un elenco di buone intenzioni. Quando il nostro Paese fa azioni contro il *dumping* sociale, ci si aspetta di essere sostenuti, come finalmente affermato inaspettatamente dal presidente Macron. Certo, ci son voluti vent'anni per arrivare alla firma ufficiale del Pilastro sociale europeo. La situazione odierna fotografa infatti un'Europa in cui i Paesi membri mantengono il controllo sulle politiche del lavoro e della previdenza sociale e nei quali è possibile vedere disparità di condizioni, disparità di salari, di pressione fiscale e di benefici tra i lavoratori dei vari Stati. Inoltre, la crisi economica ha lasciato segni profondi nelle nostre società, dall'alto tasso di disoccupazione agli alti livelli di debito pubblico, dai grandi flussi di immigrati all'incapacità di politiche atte a contingentare, regolamentare e spalmare i flussi su tutto il il continente comunitario. Tutto ciò ha alimentato anche un clima di chiusura ed euroscetticismo. Spero, signor Presidente del Consiglio, che l'adozione del Pilastro sociale europeo rappresenti una svolta fondamentale: i *leader* europei si sono assunti la responsabilità di far capire alle persone che difendere i loro diritti sociali equivale a difendere i diritti sociali dell'Unione europea, in una condizione comune di crescita e di occupazione. Per porre le basi di un'Europa sociale, occorre crederci e agire in un clima di responsabilità condivisa e azioni concrete a livello nazionale, regionale e locale, Signor Presidente, ho avuto occasione di dirlo in quest'Aula e lo ripeto: non siamo euroscettici, ma europeisti; critici sull'andamento dell'Europa, ma europeisti. Però siamo chiamati anche a essere persone di buon senso: pretendiamo, cioè, in nome degli ideali e dei principi contenuti nelle Carte europee, che si ridiscutano le politiche finanziarie e le politiche bancarie, si contrastino le nuove e le vecchie povertà e si dia senso e concretezza al Pilastro sociale europeo. Signor Presidente, a questo proposito la nostra posizione, sebbene all'interno di un Gruppo che ha diverse sensibilità culturali, può essere riassunta nelle parole dell'europarlamentare Raffaele Fitto, «Il negoziato sulla #Brexit sembra aver preso la strada giusta. Era quello che auspicavamo per cittadini #UE che che continueranno a vivere in #GB. Ma perché non cogliere questa nuova fase della vita della #UE per rivedere tutte le regole e i trattati esistenti? Perché aspettare che altri Paesi sentano il bisogno di lasciare un'istituzione che non riesce più ad interpretare il sentimento Tutto questo, signor Presidente, ci attendiamo e ci permetta di nutrire qualche dubbio sulla celerità e la convinzione con la quale il nostro Paese potrà portare sui tavoli europei queste reiterate istanze. Per tale ragione e sempre in rispetto delle grandi sensibilità presenti all'interno del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, ci permettiamo di esprimere scetticismo sulle sue odierne comunicazioni. *(Applausi dal Gruppo GAL

turistica e questa chiudendo? Questo è l'esempio di come si tutelano gli italiani? A queste persone si dà giustamente alloggio, ma i sindaci sono contrari perché gli edifici vicini subiscono inevitabilmente una penalizzazione. Perché non c'è attenzione verso gli italiani? Perché

l'accordo sulla prima fase del negoziato sulla Brexit è stato sicuramente soddisfacente, ma anche difficile. Le trattative si sono trascinate oltre quanto previsto e forse questo è dipeso anche dal fatto che spesso ci si fa trascinare nel fare scelte con la pancia, dando credito alle promesse di benefici che poi si rivelano inesistenti e scoprendo che gli svantaggi sono molto maggiori di quello che si è promesso in una campagna che è stata molto populista. Forse è stato necessario del tempo per

del popolo britannico in ordine all'uscita. Ormai è un dato fermo che la Brexit sia una scelta senza ritorno. Si tratta certamente di un divorzio non semplice, non solo per il rispetto degli impegni presi

ruolo che abbiamo sempre condiviso e che ribadiamo essere ciò che è davvero importante per l'Unione europea. Allo stesso principio è ispirata la posizione del Governo

con un Ministro dell'economia e delle finanze europeo. Sono certamente questi i punti rilevanti di una nuova fase di integrazione economica e politica. Il confronto con l'Unione europea richiede non solo regole condivise, ma anche una maggiore considerazione della condizione particolare dei singoli Stati membri. Non è, infatti, ragionevole chiedere all'Italia, che ha un debito pubblico

cento del PIL questo gigantesco debito: sono situazioni diverse ed è di tutta evidenza che non possono essere trattate allo stesso modo, applicando le stesse regole e la stessa tempistica. Sarebbe, a nostro parere, del tutto iniquo. L'Italia, negli ultimi anni, ha compiuto tantissimi sforzi, maggiori di tanti altri Paesi dell'Unione europea, e di questo, una volta tanto, dovrebbe essere essere consapevole anche l'Unione europea e chi critica spesso l'Italia. Il punto di partenza dell'Italia semplicemente era più difficile e diverso da quello Condividiamo, quindi, la posizione del Presidente del Consiglio quando afferma che la questione del *fiscal* *compact* non deve essere inserita nei trattati europei, ma deve essere oggetto di un negoziato per una direttiva europea, garantendo così la necessaria flessibilità.

rispetto a tutto quello che abbiamo sentito negli ultimi dieci anni, quando le rettifiche delle stime erano quasi sempre al ribasso, mai al rialzo. Nel nostro piccolo, come piccolo

Signor Presidente del Consiglio, la ringrazio per la relazione e per l'attenzione che ha inteso condividere con quest'Assemblea, che rinnova gli impegni e le responsabilità del nostro Paese in sede europea e che esprime coerenza rispetto al cammino intrapreso fino ad ora. Voglio soffermarmi per prima cosa su quanto è stato riferito in merito alle dinamiche della gestione della Brexit, rinnovando in questa sede l'impegno del nostro Paese, da lei ulteriormente segnalato, sul fronte della gestione dell'*impasse*, su cui l'attenzione dell'Italia è sempre stata elevata. Certamente la conclusione della prima fase dei negoziati della scorsa settimana, in cui è stato posto l'accento sui diritti dei cittadini, un segnale da ritenere positivo. Inoltre, la definizione in questo Consiglio europeo di una discussione sullo stato dei negoziati sulla Brexit e la valutazione di avviare una seconda fase dei negoziati rappresentano un passaggio particolarmente rilevante dell'intero processo. Sebbene non sia stata accolta pienamente la richiesta dell'Unione europea per quanto riguarda il riconoscimento della garanzia della giurisdizione della Corte europea sul fronte della tutela dei diritti dei cittadini residenti nel Regno Unito, ma sia stato raggiunto un compromesso in cui la Corte rappresenta comunque un riferimento per il giudizio britannico, le garanzie ottenute con l'accordo dello scorso 8 dicembre rappresentano sicuramente un passo importante. Resta il fatto che l'attenzione dell'Unione europea e dell'Italia dovrà essere elevata nel proseguire in un'azione costante di sostegno della trattativa con il Governo britannico, anche nella prospettiva di favorire l'individuazione di soluzioni che limitino le potenziali criticità *post* Brexit sui cittadini e sulle imprese. In questo la responsabilità del nostro stesso Paese deve essere determinante, anche in ragione degli impegni già contratti sul piano nazionale. infatti a quest'Assemblea il lavoro svolto negli ultimi mesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva del Comitato per le questioni degli italiani all'estero e delle Commissioni politiche dell'Unione europea, che ha condotto all'approvazione da parte di quest'Aula di una risoluzione con degli impegni molto precisi, di cui lei, Presidente, si sta facendo egregiamente rappresentante.

giusta. L'invito che verrà fatto nei prossimi giorni dall'Unione europea al Regno Unito per fare chiarezza sulla configurazione delle future relazioni da instaurare dopo la Brexit rappresenta, appunto, un approccio significativo e coerente. Merita un'attenzione particolare anche la posizione europea emersa in occasione dell'ultimo vertice sociale di Göteborg dello scorso novembre, in cui è stata sottolineata l'esigenza di mettere al primo posto le persone, focalizzando l'attenzione dunque sulle dinamiche sociali dell'Unione europea. Pertanto, tra gli obiettivi figurano quello dell'implementazione, a livello dell'Unione e degli Stati membri, del pilastro europeo dei diritti sociali e la facilitazione di un dialogo sociale efficace a tutti i livelli. Tale iniziativa si inserisce in maniera perfettamente funzionale nella prospettiva di riabilitazione dell'immagine e dell'*appeal* dell'Unione europea nel suo rapporto con la cittadinanza. Un altro tassello importante dello scenario della trattazione europea resta quello afferente alle politiche migratorie, che verranno affrontate a margine del Consiglio europeo e all'interno del calendario previsto nell'agenda dei *leader*. Una delle priorità, su cui si chiede anche nella risoluzione in esame un impegno preciso, è la revisione del Regolamento di Dublino, in coerenza con gli emendamenti avanzati di recente dal Parlamento europeo e nella prospettiva di approdare ad un sistema comune di asilo, con una normativa di riferimento chiara e uniforme, ponendo ulteriormente l'accento sull'esigenza di rinnovare l'attenzione dei *partner* europei sul fronte della gestione del fenomeno migratorio, rispetto al quale l'Italia svolge egregiamente la sua parte nel rispetto dei diritti umani e del pragmatismo, che non

Pertanto, tra gli impegni della presente risoluzione vi è anche quello di non concedere fondi europei, vincolando dunque gli «onori» dell'appartenenza all'Unione europea all'onere inderogabile del rispetto dei principi e dei valori fondanti dell'Unione europea stessa. La prospettiva a cui ci si avvia con questo Consiglio rappresenta, a mio parare, un'opportunità per rimettere in gioco le potenzialità dell'Unione e le sue priorità, in un momento in cui siamo chiamati a rinnovare i termini di responsabilità di Bruxelles. Signor Presidente, l'appuntamento europeo dei prossimi giorni assume, quindi, un carattere significativo in ragione non solo della molteplicità degli argomenti importanti in oggetto, ma anche per la delicatezza della congiuntura politico e sociale. Cito alcuni temi significativi: università europea, Erasmus plus, politiche finanziarie, difesa Comune europea, ricerca. Questo per delineare in maniera corale riflessioni e strategie sul breve e medio periodo, con l'auspicio di superare quelle incertezze che le dinamiche di compromissione del ruolo dell'Unione europea, *in primis* con la Brexit, stanno generando non solo tra i 27, ma in uno scenario globale, alle diverse concezioni dell'Europa dei 27 Paesi. Il mio Gruppo sceglie più Europa e un'Europa del futuro con identità chiara a sfidante. in ragione di tali aspetti evidenzio il voto favorevole del Gruppo Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa alla risoluzione in esame e al suo operato. *(Applausi dai

dovuto ascoltare molte volte in quest'Aula nei mesi passati, in particolare dal suo predecessore. Mi riferisco a quella propaganda elettorale anche in in tempi non sospetti, che tendeva a rappresentare un racconto del Paese molto diverso dalla realtà. Invece, presidente Gentiloni Silveri, riconosco lei ammette quanto sia profonda e stridente la crisi sociale ed economica che ha compiuto il nostro continente riconosce che il ritmo di ripresa del nostro Paese è più basso che altrove. Ciò mi sembra, rispetto a un racconto ispirato alle magnifiche sorti e progressive, che però stanno soltanto nella testa del segretario del Partito Democratico, obiettivamente un passo in avanti: è un bagno di realtà che ci pare un elemento di positivo confronto da avere in questa Aula.

come ho sentito oggi dalle sue parole, presidente Gentiloni Silveri, proprio nel giorno in cui è uscito un clamoroso rapporto di Amnesty International, onestamente stride molto con l'esigenza di un bagno di realtà. Penso che il Governo italiano dovrebbe dire delle parole chiare rispetto a quello che sta emergendo in queste ore e che peraltro alcune forze di questo Parlamento, che stanno condividendo

il nostro Governo esprimesse parole più chiare su questo punto; non possiamo accettare che ci sia un'ombra così profonda e così forte su quello che sta accadendo in Libia in questi mesi. Si parla nel rapporto di Amnesty di un sofisticato sistema di abuso e di sfruttamento di rifugiati e di migranti da parte delle autorità libiche e, soprattutto, della complicità dei Governi europei riguardo alla violazione dei diritti umani nei confronti dei migranti rimasti in Libia. I Governi europei - viene detto - sono consapevolmente complici

una fase storica caratterizzata da un rigurgito pericoloso delle forze della destra e dell'estrema destra e dal ritorno di una certa terminologia razzista, che naturalmente spaventa le anime democratiche. Chiedo allora al Governo e ai partiti di maggioranza se abbia senso manifestare in piazza contro il razzismo e, contemporaneamente, sentirsi dire da Amnesty International di chiudere gli occhi rispetto a quello che sta accadendo in Libia anche con la complicità del nostro Governo. Mi pare una domanda rispetto alla quale dovreste dire parole più nette e più chiare rispetto al silenzio assordante di queste ore. Voglio poi dire con altrettanta chiarezza, che trovo assolutamente insufficiente l'atteggiamento del nostro Governo. Mi ha colpito non sentire la parola Palestina nella relazione che il Presidente del Consiglio ha svolto pochi minuti fa.

Nella nostra risoluzione chiediamo che il Governo promuova una posizione di ferma condanna di quanto accaduto nel corso di questi giorni, che hanno visto la scellerata ipotesi del Presidente degli Stati Uniti d'America di trasferire l'ambasciata americana a Gerusalemme.

Devo poi dire che stride con tutto ciò il fatto che nel nostro Paese non si dia seguito a quello che invece il Parlamento ha voluto dire con chiarezza già alcuni anni fa quando, a larghissima maggioranza, ha votato una mozione che impegnava il Governo a farsi promotore del riconoscimento unilaterale dello Stato della Palestina. Se volete fare una cosa buona, signori del Governo, signor Presidente del Consiglio, andate al Consiglio d'Europa e chiedete il riconoscimento dello Stato della Palestina da parte dell'Unione europea. *(Applausi di mettere un punto sulla questione, di alzare una bandiera, di dire che l'Unione europea cerca di mettere in campo un'ipotesi di politica estera diversa da ciò che sta facendo l'amministrazione americana in questi anni. Abbiamo uno scenario drammatico

rispetto ad un quadro politico molto difficile e complesso, approfittando altresì di quello che la politica estera statunitense sta facendo in particolare nei confronti dell'Iran e rispetto alla questione che da molto tempo a questa parte attraversa il mondo sunnita e il mondo sciita. Ebbene, adesso è il momento di battere un colpo, di provare a mettere in campo un'ipotesi di politica estera che possa parlare a quella gran parte di mondo arabo che pure cerca una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese.

anche quella *leadership* palestinese più moderata che cerca e ha cercato in questi anni di far vivere momenti di pace, mi sembra una gravissima responsabilità politica. Vorrei che risuonassero in quest'Aula due parole, che non sono semplicemente i nomi di due Stati: Libia e Palestina, Libia e Palestina. Noi ve lo ripeteremo tutti i giorni; ve lo diremo anche quando si scioglieranno le Camere; ve lo diremo anche in campagna elettorale,

la nostra risoluzione, speriamo di poter dire - militerà sempre dalla stessa parte.

Capisco sia tardi per il Governo iniziare ad ascoltare, ma noi non ci stancheremo di fare chiarezza per dovere verso gli italiani. La prima questione sul tavolo: la via della cooperazione europea strutturata permanente in tema di difesa (Pesco), per di più solo su base volontaria, potrebbe comportare per l'Italia costi aggiuntivi rispetto alle spese militari per la difesa nazionale, per programmi che peraltro appaiono, in certa parte, complementari alla NATO. Il Gruppo Movimento 5 Stelle chiede che nel settore della difesa i programmi di cooperazione siano indirizzati a eliminare inutili duplicazioni e sprechi a standardizzare gli equipaggiamenti permettendo, quindi, economie di scala, risparmi sul bilancio della difesa negli Stati membri da reinvestire, auspicabilmente, nella lotta alla povertà, alla disoccupazione, alle diseguaglianze. Diversamente, si rischia concretamente di sovvenzionare unicamente l'industria degli armamenti. Infine, l'Unione europea deve essere protagonista nella risoluzione dei conflitti, e non invece, come troppe volte sta accedendo, parte responsabile degli stessi. Secondo tema: la Brexit. Il fragile accordo siglato sulla carta sembra una vittoria per tutti; vi si afferma il principio di non discriminazione e di parità di trattamento per i cittadini britannici in Europa e per e per gli europei nel Regno Unito, che potranno continuare a esercitare i diritti attualmente garantiti: libertà di circolazione, soggiorno, diritti sociali e ricongiungimenti familiari, che dovranno essere eventualmente interpretati dai giudici britannici secondo la giurisprudenza consolidata consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea. Eppure, i cittadini italiani - e non solo - denunciano situazioni di intolleranza e xenofobia: proprietari di case che si rifiutano di affittare a cittadini europei; datori di lavoro che pubblicizzano posti di lavoro solo per britannici; difficoltà ad aprire conti bancari e mutui e un generale "tornate al vostro Paese" rivolto ai cittadini dell'Europa dell'Est come ai giovani italiani, in particolare bambini e adolescenti. Questo deve aprire gli occhi sulle cause della Brexit: non è stata votata dalle *élite* di Londra, Oxford o Cambridge, che dalla globalizzazione hanno tratto occasione di guadagno, ma da quella parte del popolo che nelle periferie ha vissuto il massiccio ingresso di migranti dall'Est Europa come una forma di concorrenza sleale sui salari. È il sistema Europa ad apparire come un amplificatore della competizione e della conflittualità, tanto tra Paesi membri quanto tra fasce sociali; quell'Europa che il presidente Gentiloni Silveri chiamava poco fa famiglia: più volte ha parlato di famiglia europea. Ebbene, l'ultimo rapporto Censis dice testualmente: «non si è distribuito il dividendo sociale della ripresa economica».

ascolto! Dateci ascolto. Altrimenti, presto parleremo di Uexit. Sarà l'Europa a fallire dopo il fallimento di questi sciagurati Governi. Il Movimento 5 Stelle chiede che il Governo italiano si adoperi perché nelle trattative per la Brexit con le autorità britanniche si ottengano garanzie per bloccare i fenomeni xenofobi nei confronti dei nostri connazionali e degli altri cittadini europei; affinché l'iscrizione all'AIRE sia riconosciuta come elemento di certificazione della residenza in Gran Bretagna; affinché le nuove norme per l'ottenimento del certificato di residenza risultino semplici, rapide e non introducano alcuna forma di discriminazione o condizioni volte a limitare fortemente i diritti; per garantire, di concerto con le istituzioni europee e internazionali, il rispetto dei diritti umani dei migranti a seguito degli accordi conclusi con Stati terzi al fine del controllo dei flussi migratori. però, qui sospesa la responsabilità del Governo ad evitare, anche nel nostro territorio, l'aumento progressivo e inesorabile del divario tra le fasce sociali che possono e quelle che sono tagliate fuori. Se questo ha portato alla traumatica uscita di un Paese come la Gran Bretagna, che ha un tasso di disoccupazione pari al 4 per cento, potete ben immaginare quali possano essere le conseguenze in Italia, dove la disoccupazione è tripla, e il Governo è continuamente prono ai poteri forti di economia e finanza. ora al tema dell'immigrazione verso l'Europa. I Governi dell'ultimo decennio hanno gravi responsabilità nella destabilizzazione di territori cruciali ma sono stati spettatori di fronte all'aumento esponenziale degli ingressi in Italia: 40.000 nel 2013, 170.000 nel 2014, fino al 2016 oltre 180.000 arrivi Il Governo vanta come un suo merito la denuncia di questi fatti. Ma a che cosa sono dovuti questi, se non agli accordi stipulati senza alcun controllo di ciò che stava accadendo? Trentasei, infatti, sono

forme gravi di tortura, soprattutto a carico di donne e bambini; dei trattamenti inumani e degradanti; della riduzione in schiavitù. rischia di essere un ennesimo errore della politica europea sui flussi migratori e di sostenere politicamente ed economicamente milizie e *leader* a dir poco discutibili, come già abbiamo visto in Turchia. Si continua ad elargire denaro, ma non si interviene sulle cause profonde delle migrazioni e il nostro Paese è costretto a gestire un fenomeno epocale praticamente da solo. Ebbene, i partiti di Governo, con l'ipocrita astensione della Lega, hanno votato al Parlamento europeo la riforma "alla tedesca" del regolamento di Dublino: una gabbia che obbliga l'Italia gestire tutti i migranti economici da sola. Per loro non è previsto nessun riallocamento, nessuna solidarietà europea, nessuna condivisione degli oneri. Stiamo parlando di oltre 70.000 persone che devono essere rimpatriate. Ma i rimpatri sono molto difficili, visto che mancano gli accordi con la maggior parte dei Paesi di provenienza. Dunque, affare nostro. E al riguardo sono tutti d'accordo al Parlamento europeo, come qui sul Rosatellum, come sui vitalizi, come sul finanziamento ai partiti. Hanno votato sì all'ennesima truffa per gli italiani, che pagheremo a caro prezzo negli anni a venire. Poi ci vediamo recapitate le risoluzioni che dicono di andare a battere i pugni in Europa. La Lega si è accodata, per non turbare le coalizioni "a ripetere". Solo il Movimento 5 Stelle ha sempre lottato in Europa per una reale, forte e autentica solidarietà. Il principio del Paese di primo ingresso, invece, viene solo rimodulato e, di fatto, confermato. I migranti economici, a differenza dei rifugiati, rimarranno nel Paese di arrivo. Tutte le persone potenzialmente pericolose restano nel Paese di primo ingresso. E siamo lasciati soli in questo. Prima uno Stato membro diventava competente se il richiedente vi aveva soggiornato per un anno, anche se era sbarcato in un altro Paese. Con la nuova revisione non sarà più così: l'Italia, come Paese di primo approdo, sarà permanentemente responsabile dei migranti arrivati, altro che solidarietà. Il meccanismo di riallocamento non è affatto automatico: scatterà dopo le procedure dei filtri sulla sicurezza e sulla domanda. Un richiedente asilo potrà dunque essere trasferito in un altro Paese dopo molti mesi dal suo arrivo e nel frattempo sarà sempre l'Italia a farsene carico. Fra i criteri per redistribuire i richiedenti asilo, non c'è il tasso di disoccupazione, restano solo quelli del PIL e della popolazione residente, così c'è il rischio di una guerra tra poveri: da una parte i rifugiati che vedono riconosciuto il diritto a restare in Italia e dall'altra i disoccupati italiani che non trovano lavoro. Infine, è concesso un periodo di tre anni di transizione per gli Stati che sono in ritardo per l'applicazione delle procedure di accoglienza. Questi Paesi sono di fatto esonerati dal meccanismo della redistribuzione. Così facendo, si legittima l'egoismo di alcuni Stati membri che si rifiutano di applicare norme comuni per il diritto di asilo e l'Italia continuerà, in questi tre anni, ad avere più migranti degli altri Paesi europei. Siamo stati i primi, signora Presidente, a denunciare il regolamento di Dublino, che che ha trasformato l'Italia nel campo profughi d'Europa. Non avrebbe senso chiedere ancora, dopo cinque anni di mancato ascolto, a questo Governo, di farsi carico dell'interesse nazionale: sarà un governo 5 Stelle a farlo, e allora si mostrerà la differenza. Signora Presidente, signori del Governo, il consesso europeo dei prossimi giorni affronterà, come di consueto, i temi del momento: le politiche migratorie, le politiche di difesa, i negoziati con la Gran Bretagna dopo la Brexit. Come di consueto, sui temi legati al fenomeno migratorio, molte chiacchiere e pochi fatti. Uno dei pochi fatti - è bene ricordarlo - lo si è ottenuto a seguito dell'azione politica di Forza Italia in Commissione difesa al Senato, che ha indotto il Governo ad assumere iniziative nei confronti delle ONG che fungevano da fattore attrattivo. A quella iniziativa sono seguiti gli impegni dell'Esecutivo

Tra i temi da affrontare c'è innanzitutto quello della stabilizzazione della Libia e la necessità, pertanto, che l'Unione europea condivida con l'Italia il peso e i costi della pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale che per il 2018 sfioreranno i cinque miliardi nel bilancio dello Stato, di cui 3,6 miliardi solo per l'accoglienza. L'impegno del nostro Paese nei confronti dell'Unione europea deve prevedere un repentino passaggio dalle parole ai fatti, attraverso il concreto sostegno ai Paesi più coinvolti nell'attuale crisi migratoria (Italia e Grecia). La previsione di una rafforzata cooperazione tra gli Stati, scaturita dagli accordi de La Valletta, al fine di facilitare il ritorno e la reintegrazione dei migranti irregolari nei Paesi di origine, rimane ancora lettera morta. Consideriamo fondamentale condizionare l'attribuzione dei fondi comunitari agli Stati membri al rispetto degli obblighi in materia di asilo, considerato che i Paesi che più si oppongono ad ospitare i migranti da ricollocare sono quelli che più beneficiano dei fondi europei. fondamentale, inoltre, continuare ad adoperarsi affinché i Paesi di partenza dell'ondata migratoria si impegnino per un maggiore controllo delle frontiere, impedendo in tal modo la partenza e il passaggio diretto verso la Libia. È necessario, quindi, proseguire l'impegno verso una piena assunzione delle proprie responsabilità da parte dei Paesi dell'area del Nord Africa (Libia e Tunisia innanzitutto) nelle operazioni di salvataggio compiute nelle aree SAR di loro competenza. fare in modo, poi, nelle opportune sedi internazionali e nell'ambito delle relazioni bilaterali, che nessuna iniziativa non coordinata possa pregiudicare l'efficacia della nostra missione, sia diplomatica che militare, in Libia. Rimane primario, dopo Malta, l'impegno dell'Unione europea nel garantire, in Libia, capacità e condizioni di accoglienza adeguate per i migranti, attraverso la costruzione di campi di accoglienza che abbiano gli standard richiesti da UNHCR e OIM. Riteniamo, altresì necessario, con riferimento alla politica estera e di difesa comune, operare un deciso spostamento dell'asse prioritario di attenzione dell'Unione europea verso l'area del Mediterraneo, in termini di cooperazione politica ed economica. Va inoltre rafforzata la politica europea di vicinato, che mira a gestire le relazioni dell'Unione europea con i Paesi vicini, meridionali e orientali, avendo come principale obiettivo quello di promuovere l'integrazione economica e la pacificazione nelle aree di conflitto. L'Europa deve poi agire nelle opportune sedi diplomatiche, nei confronti della Tunisia, affinché si impegni a fermare la nuova rotta migratoria illegale, anche in collaborazione con il nostro Paese. Di primaria importanza, altresì, è mettere in campo il massimo impegno per prevenire il probabile tentativo di rientro in Europa, anche con le ondate migratorie, dei *foreign fighter*, già impegnati nelle aree di conflitto. Valutiamo necessario, come più volte vanamente auspicato, un migliore coordinamento tra i Servizi di *intelligence*, sostenendone il finanziamento ulteriore, anche attraverso le risorse dell'Unione europea. Con riferimento alla Brexit, l'Italia deve farsi portavoce, a livello di Consiglio europeo, della necessità di analizzare le criticità che continuano ad essere espresse con riguardo alle capacità dell'Unione europea di offrire risposte efficaci alle problematiche sociali ed economiche dell'Unione. Innanzitutto, preso atto della decisione della Gran Bretagna di uscire dall'Unione europea, il compito dell'Europa deve rimanere quello di mantenere i migliori rapporti possibili

dei cittadini italiani e del Regno Unito mantenendo un principio di equità, simmetria e non discriminazione, e assicurare quindi la certezza del diritto per le persone giuridiche e per le imprese. Infine, ma non l'ultimo dei problemi, i rapporti dell'Europa con la Federazione Russa. È necessario adoperarsi una volta di più per sostenere un accordo soddisfacente tra Russia e Ucraina che consenta all'Unione europea la normalizzazione di rapporti amichevoli con un *partner* importante quale è la Federazione Russa. Insomma, signor Presidente, i temi sono tanti e articolati e ci auguriamo che nell'interesse del nostro Paese il Governo possa affrontarli in modo finalmente più concreto ed efficace di come non sia stato fino ad oggi. *(Applausi

senatrici, senatori, componenti del Governo, vorrei fare una prima considerazione, perché forse questa sarà l'ultima occasione in questa legislatura per parlare delle politiche per il Consiglio d'Europa. La considerazione è un po' ironica e un po' estetica: è cambiato lo stile; c'è una relazione migliore con il Parlamento; c'è da parte del Presidente del Consiglio uno stile adeguato al rango. Devo dire che lo stile è certamente cambiato e che lo apprezzo molto anch'io, ma ciò che è cambiato è che nel corso di questi anni si è compiuta una sequenza di azioni che hanno cambiato la situazione. Non c'è un cambiamento dello stile, ma della situazione. Soltanto due anni fa noi eravamo impegnati

L'hanno fatto le nostre Forze armate; l'ha fatto un'eroica Guardia costiera; l'hanno fatto eroicamente le popolazioni del nostro Mezzogiorno; abbiamo fatto quello che nessun altro Paese d'Europa aveva fatto. Quando eravamo a quel punto, ci siamo sentiti dire che avremmo dovuto limitare e regolare i flussi dei migranti verso il nostro Paese.

Abbiamo fatto accordi con le comunità locali e con i Paesi più arretrati della fascia sub-sahariana, abbiamo creato le condizioni per le quali

dei Paesi africani che possono avvalersi di un accordo con l'Unione europea per cercare di sostenere le proprie economie e la propria situazione.

Sono molto contento che tante forze politiche oggi ci abbiano raccontato degli allarmi di Amnesty International circa i cosiddetti centri di accoglienza in Libia. Non ricordo però questi appelli di Amnesty International quando due o tre anni fa la gente affogava in mare, noi la salvavamo e ci sentivamo dire che stavamo facendo qualcosa contro l'interesse del nostro Paese. Amnesty International c'era allora e c'è anche adesso e adesso siamo impegnati a fare in modo che le condizioni di quei centri di accoglienza

non scaricando le proprie responsabilità sui Paesi mediterranei o anche, facendo di peggio, come alcuni Paesi mediterranei fanno nei confronti di altri Paesi mediterranei. Si fa più Europa in questo Consiglio europeo. Mi dispiace tanto per gli antieuropeisti, che erano tanti fino a qualche giorno fa. Mi dispiace per loro, ma si fa più Europa, perché quando si realizza un programma di cooperazione strutturata e permanente di difesa, si fa più Europa. Su cosa l'Europa deve strutturare il proprio modo di comportarsi e la propria unitarietà, se non nell'avere una strategia comune di difesa e di approccio alle grandi questioni internazionali? Si fa più Europa perché si mettono in discussione i rapporti tra l'Unione europea e la NATO, sulla base delle indicazioni del Vertice di Bratislava. Vorrei si ricordasse soltanto qualche mese fa c'è stato il Vertice di Bratislava, che ha definito nuovi rapporti tra Unione europea e NATO. Si fa più Europa, perché si fa un'Europa più sociale.

che si crei un pilastro europeo per la protezione dei cittadini, per la crescita e l'occupazione, il fatto che si prefiguri una carta dei diritti sociali europei, mi paiono temi che "fanno Europa". Fanno Europa sul serio, non un'Europa che parla male di sé stessa, in cui ognuno trova le responsabilità proprie in quelle degli altri; un'Europa che si impegna a perseguire con determinazione i progetti concernenti il proprio futuro delineati dall'agenda dei *leader* e negli obiettivi della Carta sociale europea; a sostenere la cooperazione strutturata per la difesa; a fare una politica estera europea che metta al centro il Mediterraneo con un partenariato strategico con l'Africa e un piano di stabilizzazione dello sviluppo multilaterale, il consolidamento di un'autentica dialettica politica europea attraverso misure come l'istituzione di una circoscrizione europea, la difesa della democrazia e dello Stato di diritto in Europa, un rafforzamento degli strumenti di difesa dell'Unione. Si parlerà della necessità di rilanciare l'idea di una procura europea contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Meno Europa? Questa è Europa;

con una qualche dignità per quello che abbiamo fatto nel Mediterraneo, per quello che abbiamo fatto con l'Africa e - consentitemi di dirlo - per quello che abbiamo fatto nel nostro Paese con i risultati economici che abbiamo prodotto, con i miglioramenti che abbiamo fatto.

e che ci consentirà di chiedere cose che a noi interessano molto, come la revisione del Trattato di Dublino, di ricordare ai *partner* e alle istituzioni europee che la gestione del fenomeno migratorio non è una responsabilità di uno solo ma deve essere condivisa e che bisogna ridurre i fondi a quei Paesi europei che rifiutano le proprie quote di migranti e di fare la propria parte rispetto ai problemi dell'immigrazione. Dobbiamo affrontare anche la Brexit e in questa sede vorrei dire brevemente che è un negoziato difficile, problematico, non semplice. Il Regno Unito è un grande Paese che esce dall'Europa; forse, se dovesse rifare quel *referendum,* oggi farebbe delle scelte diverse da quelle che ha fatto qualche mese fa *(Applausi dal Gruppo

Lo vogliamo dire o no ai federalisti di casa nostra che non c'è nessuna regione federalista in Europa che, mentre non riconosce il proprio Stato, non veda nell'Europa il proprio approdo? È così per la Catalogna, per i fiamminghi, per gli scozzesi, per tutti questi. Lo vogliamo capire o no che l'Europa è contemporaneamente riconoscimento del federalismo e delle identità regionali specifiche e contemporaneamente di una nazione unica che deve essere appunto l'Europa nella quale si ritrovano anche le minoranze?

che afferma che Gerusalemme deve essere la capitale di due Paesi e quando parliamo di due Paesi, cari amici, non parliamo della Libia e della Palestina, ma di Israele e della Palestina. Deve essere la capitale di due Paesi: uno riconosciuto, qual è lo Stato di Israele, sulla base dei confini del 1967; l'altro che deve essere democratico, pluralista, deve essere rappresentante di quelle regione, come è lo Stato di Palestina. Parliamo di una cosa seria, non facciamo della propaganda. Cerchiamo di indurre il fatto che Gerusalemme ritorni a essere una città multireligiosa e di pace e non, invece, una stimolazione della degenerazione globale. *(Applausi dal

grazie, signora Presidente.

Non sfugge a nessuno - il Presidente l'ha detto - che in Italia i tassi di crescita restano, nella media, più bassi di quelli europei, il che è giusto, purché sia chiaro che essi erano inferiori da tanti anni e che oggi il divario si sta colmando sempre più rapidamente, in particolare con

poco ruolo e poche risorse per la Commissione, che invece mette a disposizione pienamente il proprio ruolo e le poche risorse; scarsa solidarietà da parte dei Paesi, con l'eccezione, che è stata segnalata, della Germania e forse, dal punto di vista solo dei fondi e non della redistribuzione, dei Paesi del gruppo Visegrad. Voglio concludere con una notazione sulla Brexit, dal momento che trovo singolare che, a segnalare la persistenza di episodi di intolleranza e xenofobia nel Regno Unito da parte dei cittadini italiani che lì risiedono, vivono, lavorano e studiano,

è avvenuto un fatto importante per uno dei simboli dell'Italia nel mondo: il riconoscimento, come patrimonio immateriale dell'UNESCO, dell'arte dei pizzaioli napoletani.

La Corea del Sud e l'UNESCO riconoscono l'arte dei pizzaioli, l'arte di fare la pizza, il simbolo del *made in Italy* nel mondo, e noi non siamo capaci di approvare un disegno di legge che riconosca la qualifica professionale di questa figura che

Guardate che se il riconoscimento della qualifica professionale del pizzaiolo avverrà in un altro Paese e non in Italia sarete responsabili di questa vergogna, dopo che l'UNESCO l'ha riconosciuta! la Germania, la Cina riconoscessero la qualifica professionale del pizzaiolo. Diamo onore a questa gente, che porta nel mondo la cultura italiana, riconosciuta anche dall'UNESCO. Facciamolo prima che scada questa legislatura e magari ci sarà una pizza per tutti. Lo dico con simpatia a 150.000 operatori del settore, che contribuiscono per il 50 per cento al fatturato della ristorazione in Italia

Si tratta di una terra molto laboriosa che, però, all'inizio del secolo scorso, ha subìto una grave emorragia di persone che sono dovute andare all'estero per lavorare. Molti si sono trasferiti in Lussemburgo, facendo molta fatica a guadagnare quelle risorse che il proprio Paese non riusciva a mettere loro a disposizione, a causa della mancanza di lavoro. La situazione è diventata paradossale, perché quando questi nostri concittadini sono rientrati in Italia, dopo una vita di lavoro trascorsa all'estero, si sono trovati negli scorsi anni (e, nel caso specifico, anche in questi mesi), ormai pensionati, ad essere sottoposti da parte dello Stato a una sorta di inquisizione, come fossero evasori fiscali. Questo perché c'è una cattiva interpretazione di una normativa che riguarda la doppia imposizione, ovvero la dichiarazione dei redditi guadagnati all'estero, piuttosto che i redditi non dichiarati, ma guadagnati all'estero. Presidente, la situazione è paradossale e io ho presentato un'interrogazione in cui si chiede al Governo di fare chiarezza, perché ci ritroviamo con persone che hanno superato abbondantemente i settant'anni che sono classificate sostanzialmente come evasori,

arrivando alla fine dell'anno a dichiarare di aver trovato i veri evasori totali, cosa che in effetti in questo caso non è. In questo modo, tra l'altro, si infligge un grave *vulnus* nei confronti di nostri concittadini che, ripeto,

Ci sono paesi come Colorno, Brescello, Boretto e Lentigione sommersi dall'acqua. Ci sono situazioni particolarmente gravi:

a criticare la giustizia del nostro Paese, imputandole le molte piaghe che effettivamente la affliggono. Ora, però, la pubblicazione di una sentenza della corte d'assise di Milano ci offre un buon motivo per sospendere per un giorno le critiche e prendere atto di una pagina straordinaria che è stata scritta in un'aula giudiziale italiana. Straordinaria, innanzitutto, è la vicenda di un gruppo di immigrati somali che in un centro di accoglienza italiano riconoscono uno dei loro aguzzini: un membro dell'organizzazione che in Africa, col pretesto di aiutarli a raggiungere l'Europa, ha organizzato il loro sequestro in diversi "*lager*" libici, dove li ha sottoposti alle sofferenze più atroci per estorcere dalle loro famiglie una sorta di riscatto, condizione per consentire loro poi di affrontare la pericolosissima traversata del Mediterraneo. Il gruppo di rifugiati a Milano blocca il connazionale, gli contesta le atrocità commesse, ma decide di non farsi giustizia da solo, bensì di denunciarlo alla polizia. un atto civilissimo e di fiducia nell'amministrazione giudiziaria del Paese che li ospita; un atto cui l'amministrazione della giustizia risponde nel modo migliore, con straordinaria competenza, efficienza e tempestività, applicando una norma del codice penale che attribuisce al giudice italiano, su richiesta del Ministro della giustizia, la giurisdizione su crimini commessi ai danni dei rifugiati, che altrimenti non avrebbero alcuna possibilità di essere perseguiti.

non solo un'indagine complessa viene portata a compimento dalla polizia giudiziaria e dalla procura, ma si svolge anche fino alla conclusione un dibattimento che pone sotto gli occhi di tutto il mondo civile e non soltanto italiano il massacro cui sono sottoposti i profughi africani nelle mani delle organizzazioni dedite - complice la polizia libica alla "gestione" e allo sfruttamento spietato del loro tragico viaggio verso le coste siciliane e calabresi. La sentenza, che condanna l'imputato per le atrocità commesse, conclude un processo il cui svolgimento è stato caratterizzato da un'altissima tensione emotiva per la drammaticità delle vicende e l'enormità delle sofferenze che l'istruttoria ha fatto rivivere nell'aula della corte d'assise di Milano. La tensione emotiva è stata determinata dalla scelta della corte di sottolineare, nel governo del processo, la considerazione di tutte le persone coinvolte non solo le parti lese, ma anche l'imputato, sua moglie e la sua figlia bambina - come persone umane, soggetti di emozioni e affetti familiari. La stampa aveva dato notizia a suo tempo della decisione della corte di offrire all'imputato, in una pausa delle udienze, il tempo e lo spazio riservato, fuori dalle sbarre, in cui incontrarsi con le due familiari. La sentenza, di oltre 100 pagine, è un vero e proprio trattato sull'inferno attraverso il quale passano gli immigranti che vengono dal cuore dell'Africa verso le coste del Mediterraneo. Credo che di ciò va dato atto a una giustizia di cui troppo spesso diciamo solo i difetti.

a Torino nella prima mattina. C'è stato sostanzialmente un ritardo su tutti i voli determinato dalla mancanza dei mezzi necessari per sghiacciare le ali. Siccome non stiamo parlando dell'aeroporto di Lampedusa dove per fortuna il ghiaccio è merce rarissima - ma di Torino pongo il tema della gestione sia dell'aeroporto,